Presidente, la ringrazio per avermi dato la parola. Sarò brevissimo, ma credo di avere il dovere di intervenire per segnalare al Senato che ieri si è occupato della vicenda Irisbus con un dibattito molto importante che ha dato un segnale di coesione nazionale, peraltro, attraverso la responsabilità di tutti i Gruppi, a partire dalla Lega fino al Gruppo di Coesione Nazionale

situazioni di tensione, che andranno verificate, e che hanno portato a conseguenze per qualche lavoratore che manifestava e che esprimeva il suo diritto al dissenso. Comunque, a maggior ragione per via del dibattito di ieri al Senato, mi sembrava quasi doveroso sul piano istituzionale partecipare a questo tavolo; mi sono pertanto recato al Ministero dello sviluppo economico dove, all'ingresso, ho trovato altri parlamentari

credo sia corretto sul piano della dignità dei parlamentari che questi non solo non abbiano trovato accesso al Ministero, perché il Ministro evidentemente ha deciso che non potevano partecipare al tavolo, in quanto dovevano partecipare solo il sindacato, il Ministro e la FIAT - e questa può essere una scelta

di correttezza e di educazione istituzionale che va evidenziata e sulla quale le chiedo formalmente di intervenire attraverso la Presidenza del Senato. Così come formalmente le chiedo di intervenire per fare in modo che il Ministro competente, cioè il Ministro dello sviluppo economico, venga al Senato a riferire sulla vicenda Irisbus, perché questo è un modo per mantenere correttamente i rapporti tra istituzioni, soprattutto quando l'istituzione parlamentare dimostra senso di responsabilità per cercare di accompagnare il Governo in una difficile trattativa. Credo sia il minimo che si possa chiedere, o che io almeno avessi il dovere di chiedere e di chiederle, scusandomi se ho interrotto il dibattito e il confronto su temi così importanti e rilevanti come quelli che stiamo per affrontare e fronteggiare. Mi fermo per evitare di fare altre riflessioni e considerazioni sulla cultura e sull'educazione istituzionale e sul problema che forse molti considerano i parlamentari ornamentali o fastidiosi, soprattutto quando tentano di rappresentare correttamente le esigenze territoriali, anche perché chi un radicamento territoriale non ce l'ha evidentemente questo ruolo e questa funzione non li capisce e non li comprende. Presidente Viespoli, la Presidenza si farà carico di segnalare il problema al Governo per la parte che riguarda le sue prime riflessioni. Per quanto riguarda invece la la Conferenza dei Capigruppo, riunitasi questa mattina, ha approvato modifiche al calendario corrente e il nuovo calendario dei lavori fino al al 29 settembre. Rimane confermato per la seduta pomeridiana di oggi il seguito del dibattito sulle comunicazioni del Ministro della giustizia sul sistema carcerario e sui problemi della giustizia. La discussione proseguirà, fino alla sua conclusione, nella seduta pomeridiana di martedì 27. Nella seduta antimeridiana di domami sarà esaminato il disegno di legge in materia di attività venatoria in ambiti territoriali diversi da quello di appartenenza. Su richiesta del Governo, la seduta di sindacato ispettivo di domani è anticipata alle ore 15. Le ratifiche di accordi internazionali e documenti della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari già previsti in calendario saranno esaminati la prossima settimana, per consentire alla Commissione esteri e alla Giunta di concludere le procedure avviate. Il calendario della prossima settimana prevede inoltre la discussione della mozione Finocchiaro sulla istituzione di una Commissione speciale per l'esame di proposte di riforma costituzionale a partire dalla seduta antimeridiana di mercoledì 28 settembre - il seguito dell'esame della relazione della Commissione di inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti nella regione Lazio e la mozione Germontani sulla normativa relativa agli alloggi di servizio per i militari.

e a pronunciarsi sulle condizioni detentive, sul potenziamento infrastrutturale, sulla rimodulazione delle pene e sulla modalità di esecuzione delle stesse. Io stesso, che mi occupo di carceri e di detenuti da oltre un ventennio, in più occasioni ho avuto modo di contribuire ad avviare un percorso di conoscenza, di approfondimento e di soluzione delle questioni riguardanti il cosiddetto pianeta carceri. Non ripeterò, dunque, quanto ho già più volte detto, ma tenterò invece d'individuare ipotesi utili ai fini della rimozione degli ostacoli che talvolta si frappongono nei confronti della piena e completa applicazione dell'articolo 27 27 della Costituzione. Dunque, non mi soffermerò oltre misura sulle attuali condizioni carcerarie italiane. Non ripeterò che, in una cella di meno di 20 metri quadrati, vivono anche non parlerò dei ritardi con i quali i reclusi vengono sottoposti agli interventi sanitari o alle visite specialistiche; non racconterò episodi, di cui sono personalmente a conoscenza e che riguardano condizioni detentive ben al di sotto della dignità umana; non dirò delle decine di suicidi e di morti sospette di reclusi, agenti di polizia penitenziaria e persino di alti dirigenti del DAP, né degli innumerevoli atti di autolesionismo che si registrano nelle carceri italiane. Onorevole Ministro, non dirò neanche della scarsa assistenza psicologica e delle altrettanto scarse azioni rieducative poste in essere nei vari istituti; non le ricorderò neanche del sovraffollamento, né farò riferimento alla grave carenza di personale, pari, come lei stesso ha confermato oggi, a quasi 6.000 unità, senza contare il ricalcolo degli organici dovuto proprio al sovraffollamento. Così come non dirò dei costi della detenzione, oscillanti tra i 120 ed i 250 euro al giorno, legati, per lo più, ad un'organizzazione piuttosto discutibile e ridondante del sistema. Non dirò nulla di tutto questo perché sono certo, onorevole Ministro, che si tratta di cose di cui lei è già perfettamente a conoscenza, come è emerso con grande chiarezza proprio questa mattina, tanto che lei ne ha parlato in Aula, e ne ha parlato in più occasioni. Non dirò nulla perché lei, signor Ministro, decidendo di voler risiedere vicino Regina Coeli, avendo già peraltro avviato una serie di visite nelle strutture, partendo proprio dalla mia Sicilia, ed avendo annunciato in più occasioni di voler agire sulla tipologia delle pene per i vari reati, e soprattutto per i cosiddetti reati minori o a minor allarme sociale, magari riferiti a soggetti non recidivi, né delinquenti abituali, ha mostrato una rassicurante (almeno per quanto mi riguarda e per quanto ci riguarda) conoscenza della situazione. Una condizione, la sua, che la colloca al di fuori dal coro degli incompetenti che parlano di carcere per sentito dire, in maniera scomposta e disarticolata, talvolta con odio emotivo o ideologico, come se un problema di questo genere potesse essere affrontato con lo stomaco piuttosto che con la testa. Parlerò invece di responsabilità e di colpa, di pigrizia penale e giudiziaria, di scarsa propensione all'assunzione di ben retribuite responsabilità, di autoreferenzialità dell'amministrazione penitenziaria, di paradossi burocratici, di rapporti tra chi ha commesso un crimine e chi lo ha subito, di attenzione dell'Unione europea e, di recente, della magistratura di sorveglianza italiana verso i diritti fondamentali della persona umana, soprattutto quando questa è reclusa, di riduzione funzionale e non orizzontale dei costi della detenzione e della organizzazione. A proposito, onorevole Ministro, almeno lei non cada nella trappola del DAP sulla cosiddetta capienza tollerabile, altrimenti le sentenze come quella recente del tribunale di sorveglianza di Lecce, in merito al tema dei minimi spazi vitali riservati ai detenuti, contribuiranno, sia pure in minima parte, a svuotare ulteriormente non le carceri, signor Ministro, ma le casse dello Stato. Ma cominciamo con la responsabilità e la colpa. Vi pare possibile e giusto che la società continui a considerarsi non responsabile dei crimini che si commettono nel suo seno? Pensiamo forse che il deviante provenga da un altro pianeta o forse non sarebbe il caso di cominciare a riflettere sul fatto che egli è nato, è cresciuto ed ha vissuto accanto a noi senza che noi magari ce ne siamo accorti? È possibile che le famiglie, tutte le famiglie, non solo quelle dei devianti, non si siano accorte di quanto stesse accadendo nell'anima, nella coscienza, nella mente di una persona sul punto di commettere un crimine o, se ne ha avuto la percezione, è giusto che abbia lasciato fare? È possibile che la stessa grave disattenzione si sia verificata tra i vicini di casa, i compagni di scuola, i compagni di lavoro, i servizi sociali degli enti locali, persino nelle parrocchie e nei centri di aggregazione? È possibile pensare che l'inclinazione verso il delitto sia del tutto sganciata dalle condizioni di vita, di lavoro, di studio o di bisogno del deviante? che una politica urbanistica fondata sulla creazione di enormi ghetti come lo Zen di Palermo, Librino di Catania o Secondigliano di Napoli abbia aumentato o diminuito il rischio di devianza? Mi chiedo se sia vero che è l'occasione che fa l'uomo ladro o il ladro che cerca l'occasione. Vogliamo provare ad evitare le analisi sommarie e gli altrettanto sommari giudizi, magari guardando un po' più in profondità le varie vicende? Mi auguro che questo dibattito serva soprattutto a raggiungere tale obiettivo, altrimenti esso costituirà l'ennesima esercitazione retorica di cui avremmo potuto fare facilmente a meno. Certo, la colpa un delitto è di chi lo commette, ma siamo certi che la responsabilità sia solo sua o non sarebbe più onesto ammettere che un poco è anche nostra e magari capire perché, dove abbiamo sbagliato, in quali fasi precedenti la commissione del delitto si è sbagliato e chi ha sbagliato? Il mio non è, né vuole essere, il maldestro tentativo di trovare qualche esimente verso il crimine o verso il criminale; è solo l'appassionato tentativo di individuare un percorso risolutivo più completo, meno superficiale e meno romanzato. Un tempo il carcere non costituiva la pena per qualsiasi delitto e neanche oggi lo è, almeno secondo il nostro ordinamento, ma allora vogliamo dedicarci, come lei ha fatto questa mattina suggerendo alcune ipotesi, a pensare che, forse, un tossicodipendente sarebbe meglio avviarlo verso una comunità di recupero, piuttosto che verso una cella? Vogliamo pensare che chi viola le leggi sul soggiorno possa essere più rapidamente allontanato dall'Italia invece che recluso?

potrebbero essere puniti in termini finanziari o in termini inibitivi, piuttosto che a spese del contribuente dentro un carcere che non rieduca affatto? E che, forse, reati minori di questo genere (e ve ne sono a decine), che producono migliaia producono migliaia di costosissime detenzioni, si possono trattare in maniera diversa? Vogliamo pensare che le attuali procedure penali innescano il meccanismo della cosiddetta porta girevole - a cui lei stesso, ha fatto riferimento questa mattina - che avvia al carcere per brevissimi periodi, spesso immotivatamente, circa 90.000 persone all'anno? La sua, signor Ministro, è stata una relazione onesta. Ricorrere Ricorrere al carcere per qualsiasi delitto, anche per i meno gravi, costituisce un drammatico esempio di quella pigrizia culturale, penitenziaria e giudiziaria a cui facevo riferimento prima, ma costituisce anche la prova provata della scarsa propensione all'assunzione di responsabilità da parte delle *équipe* di osservazione, da parte dei magistrati di sorveglianza, da parte di frettolosi PM e di pedissequi GIP. Vogliamo provare a superare questo genere di ostacoli con competenza e razionalità? Colleghi, è lecito parlare di autoreferenzialità dell'amministrazione penitenziaria quando risulta difficile capire come e perché sono morti Cucchi, Castro e tanti altri, o quando la gestione dei trasferimenti dei reclusi avviene con costosissima e disarticolata frequenza, o quando le numerose traduzioni di reclusi è costantemente preferita al più economico e agevole ricorso ai sistemi telematici per la partecipazione ai processi? È lecito parlare di risorse mal governate quando, invece di istituire un reparto penitenziario in almeno un ospedale per provincia (cosa che farebbe risparmiare moltissimo in termini di costo del personale e di costo delle prestazioni), si preferisce sorvegliare i reclusi che ne hanno bisogno in corsie comuni con evidenti disagi per essi stessi e per gli altri degenti, impegnando decine di agenti? O di questo genere di problemi ci dobbiamo accorgere solo quando si verifica, come nei giorni scorsi, qualche clamorosa evasione? È lecito parlare di sprechi quando si trasferiscono reclusi a pochi giorni dalla loro scarcerazione, cosa che purtroppo accade frequentemente? È possibile decapitare sistematicamente i vertici del DAP, costringendo i vari dirigenti apicali a ricominciare daccapo ogni volta che si registra un avvicendamento, rallentando per mesi l'attività del Dipartimento o sperando che chi arriva ne capisca un po' di più di chi lascia? È possibile tenere chiuse numerose strutture per motivi biecamente burocratici, come stava accadendo a Gela (mi auguro che le notizie che lei ha riferito questa mattina siano È possibile, in una situazione di grave carenza di personale come quella attuale, utilizzare

nelle stesse carceri? È possibile sprecare migliaia di euro per improbabili studi sul contenimento dei costi, mentre in molte carceri manca persino la carta igienica e gli assorbenti intimi? È possibile pensare al carcere come una soluzione definitiva senza pensare che esso, così come ha avuto un prima, avrà un dopo, e che questo dopo deve necessariamente essere preparato durante la detenzione, o sarà peggio del prima? È possibile non avviare un percorso di avvicinamento tra vittime e carnefici, lasciando aperte le gravi piaghe sociali provocate dal delitto, senza neanche tentare di costruire un percorso di redenzione, da una parte, e di sia pur difficile e dolorosa comprensione, dall'altra, utilizzando la detenzione come momento reale di reinserimento e di recupero di legalità? È possibile accanirsi nei confronti non tanto e non solo del recluso, quanto degli incolpevoli familiari, anch'essi, ricordiamolo sempre, detentori dei diritti spettanti a chi è padre, a chi è figlio, soprattutto se minore, a chi è moglie, eccetera? Onorevole Ministro, all'atto del suo insediamento, consapevole che lei si trova nella fortunata coincidenza di non doversi, al momento, far carico né degli errori del passato, prossimo o remoto, né delle condizioni del presente immediato, le ho fatto avere un promemoria, che spero lei abbia già avuto modo di leggere. Non ripeterò, dunque, il suo contenuto. Mi limiterò a suggerirle un metodo. Il carcere è un luogo in cui si incrociano tante esigenze, tante verità, tanti punti di vista, tanti interessi talvolta contrapposti tra loro. La sua competenza, signor Ministro, la metterà nelle condizioni di poter comprendere bene quali siano le soluzioni più equilibrate da porre in essere. Io mi permetto di indicargliene una: metta attorno ad un tavolo il mondo della giustizia penale e di sorveglianza, i rappresentanti dei lavoratori penitenziari, il mondo della sanità penitenziaria, gli enti locali, le Regioni, i Garanti, in quanto rappresentanti dei diritti dei detenuti, i rappresentanti dell'amministrazione penitenziaria stessa ed un gruppo di esperti; avvii un confronto aperto, senza difese di parte e non autoreferenziale tra queste componenti, e vedrà che su molti temi non sarà difficile trovare un'intesa. La sua conoscenza della materia, come dicevo, farà il resto.

e in cui i dettati costituzionali non siano un mero auspicio, ma una pratica quotidiana. Sogno un Paese in cui l'unico lavoro offerto ad un recluso riabilitato non sia quello proposto da aziende di comodo e dove il mondo dell'imprenditoria sappia, generosamente, fare la sua parte. Sogno un Paese dove non si pensi al carcere come un luogo in cui nascondere gli errori della società, ma in cui si possa costruire un sistema in grado di non ripeterli. Sogno un Paese in grado di non tenere ammassate decine di persone in celle anguste e vecchie, condannandosi e facendosi condannare dalla magistratura propria ed europea per trattamenti inumani e degradanti. Sogno un Paese che sappia far tesoro delle esperienze virtuose che vengono compiute in carcere, come nel caso della legge per l'autoimpiego in vigore in Sicilia, che ha salvato oltre 120 detenuti, mai più tornati a delinquere, con costi irrisori e con vantaggi enormi. Sogno un Paese che non si accorga che esiste un problema carceri quando si alza l'indice dei suicidi e poi se ne dimentica. Sogno un Paese in cui privazione della libertà non significhi privazione della dignità e dove le colpe e le pene dei padri non vengano scontate anche dai figli, spesso trascinati nel baratro dall'insensibilità e dal pregiudizio, anche nostri, per non parlare di quelli che, incolpevoli, vengono privati della libertà al seguito dei genitori. Onorevole Presidente del Senato, onorevole Ministro forse sarò uno che non ha smesso di sperare in un Paese diverso e migliore, forse non sarò realista, ma secondo le leggi dell'aerodinamica un calabrone non dovrebbe poter volare, ma lui non lo sa, e vola lo stesso. Buon lavoro, onorevole Ministro, io e tanti come me che si occupano di carceri sono a sua disposizione e attendono da lei qualche buona notizia; non ci faccia aspettare troppo!

rilevando l'evidente abisso che separa la realtà carceraria di oggi dal dettato costituzionale sulla funzione rieducatrice della pena e sui diritti e la dignità della persona, ho sperato che effettivamente si cominciasse a parlare in maniera seria e concreta del problema delle carceri, che in fin dei conti ci siamo riuniti questa mattina in quest'Aula perché c'è un sovraffollamento indecente delle nostre carceri che sicuramente

di alleggerire il numero dei detenuti e, dall'altra, che si prendesse anche in considerazione, e che lei ci manifestasse quale fosse il suo pensiero

che poi sono state abbandonate; cosa volesse fare sul piano penale per diminuire il numero dei processi, cioè per riformare il diritto penale sostanziale, non riducendo tutto a pene detentive, ma scegliendo la strada di depenalizzare la maggior parte dei reati che potevano essere depenalizzati con una politica di di penalizzazione diversa, ma altrettanto efficace, di determinati comportamenti illeciti.

che lei non ci ha spiegato. Ha detto che è aumentato il numero dei posti in carcere di 440 unità, ma non ci ha detto perché le carceri, carceri, costruite spendendo fior di milioni di euro, non siano state messe in funzione, cioè perché mancano gli agenti carcerari. Infatti, si dice ne manchino 6.000, come ricordava anche il senatore Fleres. Tutto questo non ce l'ha precisato. C'è stata una grande delusione quando ha detto in un momento in cui bisogna affrontare il problema del sovraffollamento delle carceri, ci sono ancora disponibili 2.000 posti. Lei ha fatto una distinzione

siamo a 67.000, ce ne possono stare ancora 2.000. Noi ci aspettavamo che lei ci venisse a dire che cosa ha intenzione di fare per diminuire il numero dei detenuti

Per la verità, il problema degli stranieri c'è sempre stato. Adesso saranno il 36 per cento invece del 33 per cento, ma gli stranieri ci sono sempre stati. Signor Ministro, non è possibile fare, come ha fatto lei, una distinzione sul

Ma se i detenuti fino a tre giorni sono 21.063, non le viene in mente che questi non sono detenuti per abuso della carcerazione preventiva da parte della magistratura, ma perché sono stati arrestati e, al momento della convalida dell'arresto, che avviene appunto nei tre giorni, l'arresto sia stato convalidato, ma il magistrato non abbia emesso la misura cautelare in carcere? Questa è la spiegazione più logica. Quindi, se c'è un abuso della carcerazione preventiva, evidentemente c'è da parte della polizia giudiziaria.

che scontano una pena di soli sette giorni perché sono proprio i sette giorni che si chiedono quando si procede con il rito direttissimo e si

sempre, ed è stata risolta. E quello che mi stupisce è che non si risolva attualmente perché, tra questi detenuti, oltre il 30 per cento è tossicodipendente, la maggior parte dei quali sono piccoli spacciatori tossicodipendenti che vengono arrestati periodicamente dalla polizia e che finiscono con il riempire le carceri.

Sia nella passata che in questa legislatura io personalmente ho proposto di abolire la carcerazione per chi non commette nessun reato. degli extracomunitari ai quali non viene rinnovato il permesso di soggiorno e per questa ragione viene loro intimato di tornare all'estero. Se questa intimazione non viene eseguita, è prevista la pena da uno a quattro anni.

Quali misure alternative ci vengono proposte dal Ministro per alleggerire la posizione dei detenuti? Nessuna misura quindi, nessuna depenalizzazione, nessuna misura alternativa.

Ministro, di cui conosciamo le alte capacità, che venissero avanzate delle proposte, e che queste venissero discusse in quest'Aula, con le proposte alternative formulate dall'opposizione. Tutto questo

Signor Presidente, l'informazione che ci ha dato relativamente alle deliberazioni della Conferenza dei Capigruppo mi impone una riflessione in merito alla parte dell'odierno ordine del giorno scritta tra parentesi. Dopo aver evidenziato, in neretto, che si tratta di comunicazioni del Ministro della giustizia sul sistema carcerario e sui problemi della giustizia, nella parentesi si legge: «Come da richiesta avanzata, ai sensi dell'articolo 62, secondo comma, della Costituzione, dai senatori Bonino ed altri». Gli altri sono 140 senatori, e sarebbero stati 146 se fossimo riusciti ad ottenere anche la firma autografa di chi non era fisicamente presente due settimane fa in Senato (colgo in ogni caso l'occasione per ringraziarli). Costituzione? Dice che: «Ciascuna Camera può essere convocata in via straordinaria per iniziativa del suo Presidente o del Presidente della Repubblica o di un terzo dei suoi componenti», che è stato ampiamente superato. L'articolo 52 del nostro

il documento sul quale abbiamo raccolto le sottoscrizioni - chiaramente l'orientamento politico e anche la condivisione del documento varia, ma di così poco da averci comunque dato la possibilità di raccogliere 141 sottoscrizioni - dice che i i firmatari convocano in seduta straordinaria il Senato della Repubblica con all'ordine del giorno l'urgente discussione e votazione di un documento che fissi modi e tempi certi per l'esame di provvedimenti di amnistia, indulto, depenalizzazione e decarcerizzazione, capaci di confermare, integrare, perfezionare e rafforzare i risultati certi del progetto di riforma strutturale e funzionale della giustizia,

del Ministro stamani, dall'esordio alla conclusione, è l'anatomia di un vero e proprio delitto. Il Ministro ha omesso di dire, ma è emerso più volte nel dibattito, che per questo delitto, per questo comportamento delinquenziale della nostra Repubblica (non da ieri né dall'altro ieri, ma ormai da quasi tre decenni), la Corte europea dei diritti umani ha emesso oltre 1000 sentenze, affrontando tutte le criticità dell'amministrazione della giustizia italiana, e non soffermandosi esclusivamente su ciò che attiene al pianeta carcerario. ciò che non è emerso in nessuno degli interventi - nemmeno nelle lunghe liste, retoricamente ben articolate, buon'ultima quella del senatore Fleres, che ha fatto la disamina di tutto ciò che non avrebbe voluto ricordare, dimenticandosi magari in questo non voler ricordare la penuria

riferendomi ai poteri dello Stato (legislativo, esecutivo e giudiziario), ma soprattutto alle vittime di questa sistematica e continuata violazione dei diritti umani. Un altro dato che purtroppo non è emerso

molto minori che stanno portando finalmente a processo persone che sono ritenute essersi macchiate di crimini contro l'umanità. Insiste quindi, e si aggrava, la sistematica violazione dei nostri diritti costituzionali, che si ampliano dall'amministrazione della giustizia, e quindi anche relativamente al pianeta carcere, a ben altro. Sono cinque mesi che, a fasi alterne e molto rallentate, Camera e Senato mantengono la Consulta senza un giudice e il Consiglio superiore della magistratura senza un membro. Anche questa è una violazione della nostra Costituzione.

Siamo chiamati spesso a votare su provvedimenti, buona ultima la manovra finanziaria, senza poter affrontare nel dettaglio le questioni, ma con il ricorso sistematico alla fiducia,

che hanno mandato in Parlamento - giocando a volte una sorta di terno al lotto, perché le liste sono bloccate - i loro rappresentanti.

e non credo che manchino né da parte della maggioranza né dell'opposizione proposte che vadano in questo senso. Anzi, salutiamo la creazione di un comitato di esperti da parte del Ministro stesso che proprio di questo dovrà discutere nelle prossime ore. Tuttavia, la riforma della giustizia magari sarebbe stato meglio farla per legge ordinaria, piuttosto che per modifica costituzionale del nostro ordinamento giudiziario - ma occorre farla dopo che abbiamo preso una decisione di vera vera e propria amnistia. Il senatore Li Gotti, nel suo dotto e articolato intervento, ha parlato dell'unghia sporca, senza però soffermarsi su ciò che quel dito, che abbiamo voluto puntare contro una luna sempre più sporca e inquinata, rappresentava con la raccolta delle firme. Forse non è un caso che nessuno dei Gruppi dell'Italia dei Valori o della Lega Nord abbia sottoscritto la richiesta di convocazione straordinaria. Egli ha detto se l'indulto svuota le carceri, l'amnistia svuota i cassetti. Noi riteniamo che carceri e cassetti (per cassetti intendiamo quelli dei nostri tribunali) debbano essere svuotati. Sicuramente è un provvedimento che, se raccontato nei termini in cui viene raccontato da chi ha votato per l'indulto, ma poi è andato a fare autocritica a reti unificate (penso sempre all'onorevole Di sicuramente risulta un provvedimento impopolare. Se invece lo si potesse articolare in tutta la sua problematicità - mi riferisco a quei *cahiers de doléances* (che ricordava fin nel minimo dettaglio poco fa il senatore Fleres) di che cosa noi imponiamo a detenuti, polizia penitenziaria, direttori e familiari degli stessi - molto probabilmente il consenso popolare aumenterebbe. Occorre quindi passare speditamente, in prima battuta, entro la giornata di martedì, a modificare l'ordine del giorno. Quest'ultimo è il frutto di un'iniziativa parlamentare - pensate voi - di un Parlamento di nominati che ha trovato la dignità individuale di 141 senatori e di oltre 250 deputati di proporre al dibattito interno dell'organo legislativo misure che affrontino, con date e tempi certi, questioni relative all'amnistia, all'indulto, alla decarcerizzazione

da questo sussulto di dignità di un Parlamento di nominati non può uscire un ulteriore rinvio alle calende greche o all'uso di condizionali che ha caratterizzato - purtroppo - la conclusione dell'intervento dell'onorevole Ministro. Occorre prendere il toro per le corna e lo si può fare esclusivamente con un provvedimento di amnistia. Se poi tra gli amnistiati ci dovesse rientrare anche il Presidente del Consiglio,

e quindi assumere questa gravissima, ma altrettanto necessaria e urgente decisione (verrebbe da dire obbligatoria, se dovessimo dare seguito ai vincoli internazionali che la Repubblica italiana ha), passando immediatamente all'amnistia. Occorre quindi modificare l'ordine del giorno e fare martedì un dibattito che passi

che anche la maggioranza ha detto di mettere al centro della necessità della riforma della giustizia: separazione delle carriere, magari anche abolizione dell'obbligatorietà dell'azione penale, che non così erano articolate nel disegno di legge uscito dal Consiglio dei ministri. Vi

Ed è sicuramente una discussione che, intanto, deve rispondere a una duplice esigenza. Infatti, da un lato, c'è un'aspettativa tra addetti ai lavori e detenuti, tendente a capire quali indirizzi saranno accolti da Governo e istituzioni per affrontare una situazione oggettivamente - come da lei riconosciuto - fuori dalla normalità e, dall'altro, c'è, più di sfondo ma fortemente condizionante, il giudizio dell'opinione pubblica e, in definitiva, degli elettori sulle posizioni che ciascuna forza politica tenderà ad assumere. Consapevoli di questo prestiamo la dovuta attenzione alle posizioni più radicali che emergono nel confronto ma non le riteniamo condizionanti. Dal nostro punto di vista, anzi, pensiamo che non ci porterà molto lontano affrontare la situazione delle carceri con il *cliché* della faccia feroce o con la semplice richiesta di una sorta di amnistia strutturale periodica. Conosciamo tutti alcuni dati, quelli che lei ci ha fornito, e sostanzialmente ci portano a dire che l'Italia è il Paese europeo che ha avuto l'aumento più consistente di popolazione carceraria dal 2007 ad oggi. Di fatto, ci troviamo, rispetto alla capienza regolamentare, con un terzo di detenuti in più. Purtroppo, all'aumento della popolazione carceraria non ha fatto da contraltare un conseguente aumento degli addetti alla Polizia penitenziaria. Secondo i dati che lei ci ha fornito - alcuni sindacati me lo dicono - - servirebbero almeno altri 8.000 agenti, considerato il sistema di turnazione che hanno, per non parlare della quantità esigua di educatori e psicologi. Se guardiamo fuori dai nostri confini, l'Italia presenta una densità penitenziaria del 153 per cento, seconda solo - come lei sa - alla Bulgaria. Il resto dell'Europa è tutta entro i limiti di tollerabilità. Inoltre è da record la percentuale di detenuti in attesa di giudizio, come le lo è la stessa percentuale di detenuti stranieri, che è molto superiore alla media europea. Siamo un caso unico che ha il triste primato del peggiore sistema penitenziario in Europa. L'analisi dei dati regionali ci dice che spetta alla Puglia il triste primato: ogni 100 posti vi sarebbero 88 detenuti in esubero. Ma in Emilia-Romagna l'eccedenza è pari a 83 unità. Come dire che questo è un problema che unisce l'Italia senza alcuna differenza geografica. Se si guarda poi alla composizione della popolazione carceraria si ritrova che un terzo è composta da detenuti stranieri: è improbabile pensare che nel prossimo futuro l'immigrazione rallenti, ed è da illusi non voler fare i conti con il fatto che le due curve immigrazione e popolazione carceraria - evolveranno insieme. Un altro terzo dei detenuti - come ci ha detto - è costituito da tossicodipendenti che, insieme agli psichiatrici e agli autori dei cosiddetti reati di strada, rappresentano le categorie più comuni. Oltre i due terzi quindi della popolazione carceraria si colloca in una fascia di disagio socio-economico e psichico. È come se ci trovassimo di fronte ad una sorta di detenzione a sfondo sociale che finisce per svolgere una funzione atipica, quasi di riduzione del disagio, delegandolo alla gestione dell'istituto della carcerazione. Un ultimo dato riguarda le circa 30.000 persone detenute in attesa di giudizio che, insieme alla cifra indicibile degli anni di detenzione inflitti ma mai scontati, rappresenta un'altra anomalia unica e insostenibile. Le previsioni prossime non ci fanno stare tranquilli. Si stima che, nel giugno 2012, la popolazione carceraria potrebbe sfiorare quota 100.000 unità. Il sovraffollamento comporta la situazione che sappiamo, in cui un detenuto si trova costretto a vivere, mediamente, con altre tre persone, in meno di 4 metri quadri *pro capite*, rispetto ai 7 fissati dal Comitato per la prevenzione della tortura, istituito dal Consiglio d'Europa. Ricapitolando, dopo cinque anni dall'ultimo provvedimento svuota-carceri la situazione è di un terzo in più di detenuti, con migliaia di agenti in meno di quelli necessari, in poco più della metà rispetto agli spazi previsti dal Consiglio d'Europa. Alla luce di questi numeri, non ci meraviglia che l'Italia sia stata condannata dalla Corte europea dei diritti dell'uomo. A rafforzare tali orientamenti cito anch'io la recente ed emblematica decisione di un magistrato di sorveglianza di Lecce che, per la prima volta in Italia, ha riconosciuto a un detenuto il risarcimento del danno esistenziale per la violazione di spazi minimi entro i quali scontare la pena. Se queste sono le condizioni, non ci si può meravigliare delle reazioni, talvolta estreme, da parte dei carcerati: è significativa la relazione tra il tasso di sovraffollamento e il numero di persone che hanno deciso di togliersi la vita in carcere. Da Da tale quadro emerge però la necessità di agire con un ventaglio di misure, strutturate e non emergenziali, in grado di razionalizzare il sistema detentivo italiano. L'indicazione fondamentale, che deve sostenere l'azione complessiva di risanamento della condizione carceraria in Italia, è il fin troppo citato articolo 27 della Costituzione, laddove recita che: «Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato». È lo stesso Presidente della Repubblica che ce lo ricorda, come lei ha sottolineato all'inizio del suo intervento. C'è dunque la necessità di risolvere il problema, ineludibile ed urgente, degli spazi, che va affrontato in modo ragionato e strutturale. Le contingenti esigenze di bilancio sono estremamente severe, ma ciò non deve e non può costituire alcun alibi. Anzi, questa condizione deve stimolare lo studio di misure innovative, sul modello del *project financing*, del *leasing*, della permuta e di tutti gli altri strumenti finanziari utili per coinvolgere capitali privati nella realizzazione e gestione di nuove residenze carcerarie. Ad esempio, in merito al *project financing*, per le residenze con livello di sicurezza basso o ordinario, che lei stesso ha citato, si potrebbero ipotizzare meccanismi in grado di collegare il ritorno atteso del finanziamento con i redditi derivanti dalle attività lavorative esercitate negli istituti, per intenderci sul modello già operante delle comunità terapeutiche. Per quanto riguarda poi la permuta, si potrebbero anche utilizzare alcune di quelle ormai famose strutture, incluse le pertinenze demaniali, già realizzate ma mai entrate in funzione a causa dell'elevato ulteriore costo che comporterebbe una loro messa in esercizio. Connesso al problema della disponibilità degli spazi è il principio della rieducazione del condannato, sancito solennemente dalla nostra Costituzione. Da molti, e nel comune sentire, detenzione è sinonimo crudo di scontare la pena. Nulla di più, e in tale via il dettato costituzionale è stato derubricato a mera norma di principio. Occorre, al contrario, dare attuazione al principio secondo il quale il periodo della espiazione della pena deve tendere alla rieducazione del condannato. Il rispetto di tale precetto resta fondamentale perché, e non è un caso, esso è previsto nel Titolo relativo ai rapporti civili della nostra Carta fondamentale. La rieducazione del condannato è un lungo percorso, che deve maturare nelle strutture carcerarie con il contributo di tutti gli operatori. La stessa promozione del lavoro nelle carceri deve essere sostenuta attraverso apposite risorse. L'inserimento lavorativo è una dimensione estremamente importante, poiché da essa - e le stime lo confermano - derivano significativi risultati anche in termini di prevenzione della recidiva. Anche se il dopo fosse il «fine pena: mai» - e molti di noi osteggiano quest'idea - siamo dell'idea che la civiltà di un Paese si misura anche dalla sua capacità di non abbandonare nessuno al proprio destino. Questo è un canone di civiltà assoluto che non ammette deroghe e, anzi, impone ogni sforzo in vista della sua attuazione. Se la pena deve tendere alla rieducazione del condannato, e la rieducazione è un processo cognitivo ed educativo articolato ed assistito da specifiche professionalità, ne deriva una nostra contrarietà a provvedimenti di clemenza generale spesso intesi come soluzione ideologica del problema. Il processo di rieducazione insito nel concetto di pena deve fornire gli elementi per supportare, o quanto meno tentare, un possibile progetto di vita per il dopo pena, rispetto al quale un'interruzione generalizzata rischierebbe di far venir meno alla radice il ruolo di guida di tale processo, peraltro costituzionalmente previsto. Sia chiaro: alcuni di noi hanno votato nella scorsa legislatura l'indulto, ed io mi iscrivo al partito di quanti, nelle condizioni date di allora, lo rifarebbero, nonostante abbia verificato che nell'opinione pubblica vi è stata una percezione prevalentemente negativa del provvedimento, al punto da farlo apparire come una scelta fortemente impopolare. Sapevamo già allora che aveva ragione chi ci segnalava un prezzo da pagare, sul piano morale e politico, non appena qualcuno dei beneficiari sarebbe tornato a delinquere, così come eravamo consapevoli che si sarebbe solo rinviato il problema del sovraffollamento carcerario, ma molti di noi votarono quel provvedimento per ragioni politiche e culturali. L'ultimo indulto era stato concesso nel 1989, tanti anni prima, ben diciassette, e dal 1992, con legge costituzionale, è stata prevista una maggioranza dei due terzi dei componenti delle Assemblee per concederlo, così come per l'amnistia. Eravamo allora, in sostanza, a ridosso della fine della cosiddetta prima Repubblica, cadeva il Muro di Berlino. La legge costituzionale sull'indulto si riformava di conseguenza. Finivano i tempi degli indulti e delle amnistie concesse con una certa frequenza, alcune delle quali, non facciamo fatica ad ammetterlo, di grande valore storico e politico, come ad esempio quella concessa su iniziativa di Togliatti. Ma oggi non ci troviamo di fronte all'ipotesi di un provvedimento di clemenza generale di quella natura, anche perché nessuno potrà mai convincerci che esista la necessità di amnistiare un gruppo dirigente complessivamente. Forse lo si potrebbe utilizzare per offrire un salvacondotto a qualcuno; parliamone, ma una discussione siffatta non riguarda lontanamente il problema del sovraffollamento delle carceri. Alcuni di noi sono invece consapevoli che questo è un Paese che ha una sua coscienza vera delle carceri e della questione dei detenuti, non solo come frutto di un'antica impostazione di sinistra, quella che riteneva le carceri come particolare strumento di lotta di classe, ma, per esempio, quella che si richiama all'ispirazione cristiana, ricordata da Giovanni Paolo II nel suo famoso discorso alle Camere congiunte. L'applauso conseguente di allora, non tanto il discorso in sé, rappresentò un impegno e un obbligo per il Parlamento; obbligo mantenuto a dimostrazione che le carceri testimoniano per alcuni la sofferenza e il limite della città dell'uomo. Non è un caso che da sempre carceri e ospedali siano state costruite nel centro delle città, per impedire che sia dimenticato che esistono luoghi della sofferenza e del dolore. Occuparsi degli infermi e dei carcerati era ed è un obbligo per chi si richiama ad alcune ispirazioni. Per dirla con altre parole, siamo consapevoli che la privazione della libertà che la società con le sue regole sancisce riguarda tutti noi e non solo i detenuti. Nello specifico però nutriamo serissimi dubbi che con un'amnistia da concedere dopo solo cinque anni dall'ultimo provvedimento svuota-carceri si possa inverare il dettato costituzionale. Ancora una volta si tratterebbe di posporre il problema, che è quello di pensare ed immaginare una riforma strutturale del sistema, reperire i fondi necessari, riformare il sistema giudiziario oltre che garantire, giustamente, la sicurezza di "Abele". Ovviamente, sappiamo bene che c'è una discussione di fondo da approfondire sul tema della detenzione e del sovraffollamento carcerario, che spazia dai contenuti della bozza Pisapia in merito alla cura in luoghi diversi del carcere per i tossicodipendenti, fino ad arrivare all'introduzione del cosiddetto numero chiuso: se lo Stato è in condizione di recludere un numero limitato di detenuti deve rispettare quel limite fino a che non ha creato le condizioni per una capienza maggiore. Così come sappiamo che c'è una interessante discussione sulla legittimità dell'uso delle carceri, e quindi della stessa modalità di espiazione della pena, per qualsiasi tipo di reato, anche quelli profondamente diversi tra di loro. Sappiamo però che, a prescindere dal tipo di approfondimento o di approccio, tutte le impostazioni che si occupano del sovraffollamento carcerario partono dal presupposto di ritenere inammissibili alcuni eccessi, come, ad esempio, come lei ci ha ricordato, signor Ministro, la constatazione che con oltre il 40 per cento di detenuti in attesa di giudizio si continua a fare un uso così sconsiderato della carcerazione preventiva, che dovrebbe essere invece l'*extrema ratio*, da adottare quando tutte le altre ipotesi alternative non sono ragionevolmente possibili, prima fra tutte la detenzione domiciliare. È proprio tornando a ragionare in chiave deflattiva sulla densità della popolazione carceraria, mantenendo fermi il principio e le finalità rieducative della pena, che sarebbe utile porre un'adeguata attenzione al complesso delle misure alternative alla detenzione. In questo senso, i dati dell'amministrazione penitenziaria a noi sono di conforto. Il detenuto cui viene concessa una misura alternativa al carcere ha una recidività minore rispetto a chi sconta la propria pena all'interno di una cella: la recidiva, trascorsi sette anni dalla pena, si attesta intorno al 19 per cento in caso di pena alternativa, mentre raggiunge il 68,4 quando la stessa viene eseguita in carcere. Per questo noi pensiamo e proponiamo di potenziare misure quali il lavoro di pubblica utilità, la detenzione domiciliare, l'ampliamento dell'affidamento in prova e così via, avvalendosi, con le opportune cautele, di strumenti elettronici di controllo della persona

Se qualcuno ha sbagliato, il Ministro e gli organi di competenza sapranno dirci dove sono finite le risorse in questa tecnologia. Ma è strano che questa sia una tecnologia che nel nostro Paese non si può adottare. proprio il braccialetto elettronico, come emblema della tecnologia che si dovrà applicare per la sicurezza anche nel campo dell'espiazione della pena. Faccio un esempio concreto, così da capirci con il signor citando l'articolo 14 dell'ordinamento penitenziario che specifica come «il numero dei detenuti e degli internati negli istituti e nelle sezioni deve essere limitato e, comunque, tale da favorire l'individualizzazione del trattamento». Con i numeri citati su detenuti e agenti, signor Ministro, questo articolo e tutta l'impostazione della sicurezza all'interno degli istituti di pena, non è più applicabile. Il vecchio sistema di controllo individuale, del tipo «uomo a uomo», è da tempo fuori dalla discrezionalità dell'amministrazione penitenziaria. Bisogna riformare completamente il sistema. Non si può più applicare il vecchio metodo del secolo scorso agli istituti carcerari e al confronto fra agenti penitenziari e detenuti. Se non si riforma profondamente anche questo aspetto e si innova investendo in tecnologia della sicurezza, nella progettazione, addirittura nell'architettura, nella costruzione e nella gestione stessa delle carceri, molte risorse rischiano di essere quanto meno mal utilizzate, se non addirittura sprecate. signor Ministro, noi abbiamo apprezzato alcune delle sue proposte. Se è interessato, vorremmo approfondire e aiutarla nel proporre qualche provvedimento come quello sulle traduzioni. Bisogna, però, ridurre il rapporto che esiste fra agenti e detenuti, senza fare scadere il coefficiente di sicurezza che deve esistere all'interno delle carceri. Ed è solo con le nuove tecnologie che potrà ottenere questo obiettivo. In ultimo, alla definizione di un rinnovato assetto del sistema carcerario contribuirebbe, a nostro avviso, l'adozione di un Garante nazionale per i diritti delle persone detenute, quale organo di vigilanza sul rispetto dei princìpi di umanità e di rieducazione della pena come sopra declinati, che si muova anche con il compito di contribuire a realizzare una rete operativa di Garanti regionali e locali in grado di fornire una tutela minima standard, garantita ed omogenea in tutte le realtà italiane. Sinceramente, se io fossi al posto del Ministro non lascerei la possibilità che esistano regioni e territori del nostro Paese che sono all'avanguardia rispetto a questi aspetti ed altri che, invece, si trovano molto più indietro. Il problema non è dei territori; è dei detenuti. In realtà, l'emergenza carceraria non è altro che la cornice di un quadro più ampio costituito dall'intero sistema giudiziario del nostro Paese, in questi ultimi anni sottoposto a modifiche introdotte da interessi di parte e non già da riforme organiche. Non è pensabile trattare il tema delle carceri disgiuntamente da una strutturale riforma del sistema giudiziario e da una forte depenalizzazione di alcuni reati di minor impatto sociale. Non giovano certamente i tatticismi procedurali introdotti dalle norme sul cosiddetto processo lungo che rischiano di alimentare azioni dilatorie a tutto svantaggio della ragionevole definizione dei processi e, cosa ancor più grave, non giova la miopia di un Governo, sostanzialmente limitato sul capitolo giustizia. Del resto il livello di credibilità e di affidabilità di questa compagine governativa è sotto gli occhi di tutti ed assolutamente insufficiente in tutti i settori. Ed anche per questo noi non siamo ottimisti. Signor ma come è possibile che chi l'ha preceduta in tre anni, quando vi era una maggioranza al massimo del suo splendore, con numeri mai visti nella storia della Repubblica italiana, riuscito a realizzare 440 posti e a ristrutturarne un altro migliaio? Adesso lei ci viene a dire che si prevede la costruzione entro il 2013 di 3.410 posti, prevede di ristrutturarne per lo stesso anno altri 710, c'è una procedura di gara per fare 4.000 posti entro il 2012, riunirà il comitato per le carceri di bassa sicurezza per altri 5.000 posti. Ministro, lei fa parte di un Governo che non ha più la forza per assumere questi impegni: manca di credibilità il Governo nel suo complesso, non la sua volontà. Per questo, noi non siamo ottimisti, anzi, riteniamo che anche in questa emergenza, come per tanti altri aspetti che riguardano la vita degli italiani, l'unica cosa che sarete in grado di fare è di lasciare la situazione molto peggiorata rispetto a quella che avete ereditato.

un sussulto positivo, mi è sembrato di percepire un'aria nuova, certamente uno stile nuovo, non più tagliente e forse anche un po' arrogante, politicamente parlando, come era lo stile del suo predecessore: lei è più accorto ed anche più accattivante.

la delusione, perché lei ha cominciato a descrivere la situazione, che è assai grave e drammatica (il sovraffollamento, i suicidi, il degrado), e ha tentato lo capisco, ma ormai non c'è più tempo e spazio per questi tentativi - di assicurare che qualcosa è stato fatto e che qualcosa si sta facendo, ha citato il Presidente della Repubblica (ormai è una regola per tutti), quindi ha indicato come possibili soluzioni da attuare traduzioni minori, trattenimento nelle celle di sicurezza presso i posti di polizia e riduzione della custodia cautelare. Nulla ci ha detto sul fantomatico piano carceri, almeno in termini concreti. Per motivi di tempo limiterò la mia attenzione, il mio tentativo di contributo, molto sereno, mi creda, a questi punti. Lei è persona intelligente, e non può non sapere

perché è inutile spiegarlo: abbiamo condotto in passato delle battaglie per evitare di lasciare il cittadino nelle mani delle polizie, per quanto evolute e democratiche possano essere, e lo sono, sotto molti aspetti, le nostre, perché nel momento in cui un cittadino viene arrestato non può e non deve rimanere nelle mani di chi lo arresta, ma deve essere posto in una condizione di trattenimento neutrale e garantito. Quindi, questo non è un riguarda la riduzione della custodia cautelare in carcere, lei ha avuto la buona maniera di non attribuire alla cattiveria dei magistrati l'uso abbondante o eccessivo delle custodie cautelari. signor Ministro, non può non comprendere - e sono sicuro che ne è certo - che parlare di carceri e parlare di giustizia è un tutt'uno: non possiamo affrontare il mondo e la miriade di problemi del carcere se non li affrontiamo in un contesto di vera, concreta e seria riforma della macchina giudiziaria. Le custodie cautelari vengono effettuate sulla base di norme vigenti: quindi è il Parlamento che deve assumersi la responsabilità di dire fino a che punto si può o non si può andare per la custodia cautelare. Ma c'è un altro aspetto che a me preme in questa sede sottolineare: finché avremo un'amministrazione della giustizia che a noi dice se un cittadino è responsabile o meno dopo sei, sette, otto dieci, la custodia cautelare resterà l'unico strumento che dice al Paese, anche a quella forte e diffusa aspettativa di giustizia, che c'è ancora una risposta repressiva giudiziaria. È l'unico Paese, il nostro,

governando, non trova la forza, non ha la volontà di porre fine a questo sistema? Non sono i magistrati che devono «calmarsi» rispetto alla custodia cautelare, siamo noi che dobbiamo avere la forza e la volontà politica di dare una svolta. Noi, cominciando dai singoli senatori nelle singole Commissioni. Se qualcuno invece

che non è stato fatto in questi tre anni. Abbiamo presentato disegni di legge che indicano chiaramente gli strumenti in presenza dei quali si incide decisamente anche sul numero dei detenuti. E perché non li abbiamo esaminati? Perché siamo stati costretti, talvolta giorno e notte (non è un'esagerazione), a interessarci di leggi che nulla avevano a che fare con il funzionamento della giustizia, ma erano solo leggi che servivano a qualcuno. È inutile persino ricordarlo

apro una parentesi, signor Ministro: non vuol fare qualcosa perché finalmente si vari la legge contro la tortura? Siamo veramente arretrati. Chiudo la parentesi e le dico: è possibile che lo stesso Stato poi, dinanzi ad una condanna dello Stato giustizia, taccia nel momento governativo? È un momento diverso, ma è lo Stato. Dobbiamo uscire da questo paradosso insostenibile: lo stesso Stato democratico che afferma sta praticando la tortura nelle carceri non fa nulla perché questo non accada più. Non è possibile limitarsi a dire che verranno costruite nuove carceri, che ci saranno 4.000 posti letto chissà come e quando, perché questo è un fenomeno esponenziale.

e giuridica insieme. Bene, signor Ministro: «insieme» significa mettersi intorno a un tavolo e lavorare nelle Commissioni, vedere quali sono i provvedimenti urgenti che insieme possiamo varare.

Invece assai spesso - come temo che possa accadere questa volta - si parla ad oltranza, ci si confronta, si urla, talvolta ci si accapiglia, verbalmente, e poi tutto finisce nel nulla. Temo a tal proposito che l'amnistia, se non inquadrata al momento giusto e nell'ambito di un sistema, di un accordo, e di un avvio concreto di riforme farebbe la fine delle altre amnistie, colleghi, amici rispettabili (io rispetto moltissimo gli amici del Partito Radicale). L'amnistia non può restare ciò che è stato nel passato, e cioè un salasso (in passato si curavano le malattie gravi con il salasso), senza servire a nulla, assoluta, perché nello spazio di poco tempo si riempiono le carceri, con una reazione sul piano civile e del discredito delle istituzioni. Non possiamo restare fermi; deve iniziare un programma che incida realmente sull'ingresso nelle carceri italiane; dobbiamo fermare questo flusso. Signor Ministro, noi possiamo farlo. Non so quanto tempo avremo a disposizione nella legislatura; temo che potremo averne poco, ma, per il tempo che abbiamo, tentiamo di fare qualcosa di concreto. Smettiamo di dire tutti insieme che la situazione nelle carceri è grave e insostenibile, perché questo ormai lo sanno tutti: noi dobbiamo dare una risposta ed evitare di fermarci solo alle discussioni.

ma sono fatti noti, provvedimenti urgenti, incisivi, concreti e seri; se ne adottiamo almeno alcuni daremo una risposta, altrimenti avremo fatto un ennesimo inutile parlare tra di noi.

da una gran voglia di lavorare, da capacità o - spesso - desiderio di integrazione. Nel corso degli anni i risultati si sono tradotti in un incremento esponenziale della criminalità e quindi della popolazione carceraria.

il 50 per cento è in attesa di giudizio, mentre il 46 per cento sconta una pena definitiva e ciò significa che nel nostro Paese è più facile scontare una misura di custodia cautelare preventiva in carcere che una pena definitiva. Chiaramente, al di là dei dati, dobbiamo porci anche delle domande: quali sono le soluzioni a tutto questo? Il ministro Maroni parlava di rimpatrio dei detenuti stranieri, che lui ha già proposto e sottolineato. A tale riguardo disse e dice che ci sono degli accordi bilaterali con i Paesi stranieri ed è questa la strada che il Governo dovrebbe seguire affinché i detenuti scontino la pena nei loro Paesi d'origine. Mi sembra una proposta di buon senso. Maroni ha osservato che abbiamo già due accordi: uno con la Romania e l'altro con l'Albania; stiamo lavorando per garantire la loro applicazione, a patto che anche in questo caso vi sia la massima sicurezza, perché se questa non c'è allora è meglio che i detenuti stiano in carcere qui piuttosto che siano liberi in Europa, come dice sempre il ministro Maroni. Chiaramente, il concetto che deve prevalere è sempre quello secondo cui chi sbaglia paga. Chi sbaglia deve giustamente espiare interamente la propria pena per risarcire la comunità danneggiata dal proprio comportamento delittuoso. Noi della Lega Nord condividiamo la funzione rieducativa della detenzione carceraria, ma spesso quest'ultima prende purtroppo il sopravvento sulla funzione rieducativa.

ha veramente ragione. Proviamo solo a pensare a quanti lavori manuali queste persone, questi detenuti potrebbero fare. Per esempio, scendendo nei scendendo nei particolari, pensiamo a quanta erba abbiamo da tagliare lungo i fossi o i bordi delle nostre strade, a quanti rifiuti da raccogliere, magari in quel di Napoli,

è sempre lo stesso: mancano i soldi per la manutenzione; non ci sono risorse. Ma perché non ci mandiamo i detenuti meno pericolosi a pulire gli alvei dei fiumi? Questo vuol essere solo uno spunto, un momento di riflessione. Ma perché gli ultimi due o tre anni di detenzione, la cosiddetta pena residuale, non li facciamo scontare pulendo i boschi e prevenendo quindi le frane? Tante sono le potenzialità lavorative di queste persone. Iniziamo a capire e a ragionare su come fare per poterle utilizzare in modo utile. Svuotiamo parte delle carceri, rispettiamo la funzione rieducativa e, sopratutto, risparmiamo denaro. ogni detenuto in carcere costa allo Stato in media 150 euro al giorno; se moltiplichiamo questa cifra per i circa 68.000 detenuti, scopriamo che il nostro Paese deve spendere oltre 10 milioni di euro al giorno per i detenuti in carcere. Le criticità delle carceri italiane sono ormai note a tutti, hanno raggiunto un livello di cronicità ormai drammatico e di sicuro vanno pertanto affrontate in modo strutturale, senza demagogia, senza strumentalizzazioni, ma, soprattutto, senza atti di buonismo ingiustificato. La storia recente ci insegna che il problema del sovraffollamento delle carceri non può essere affrontato e risolto a colpi di indulto. Gli indulti, gli atti di clemenza generalizzati e le amnistie sono stati un errore, un'indecenza politica e un totale fallimento operativo.

ha decretato, senza se e senza ma, il totale fallimento dell'indulto. Infatti, più di un terzo dei detenuti che hanno beneficiato di questo provvedimento sono incorsi nella recidività del reato, tornando pertanto a delinquere e a occupare nuovamente le patrie galere. Oggi siamo ritornati a un numero di carcerati superiore al numero di prima dell'indulto. Ci sono più carcerati in carcere oggi che prima dell'indulto stesso. Infatti, l'indulto ha rappresentato una resa incondizionata della comunità, della collettività e dello Stato nei confronti dell'individuo. L'indulto è stato chiaramente un errore politico, una beffa per tutti i cittadini onesti e per tutte le vittime di reati, anche particolarmente odiosi e gravi, purtroppo, che ha visto solo il Gruppo della Lega Nord votare contro e opporsi con forza all'entrata in vigore della legge stessa. Quindi non solo l'indulto non ha risolto il problema del sovraffollamento delle carceri, ma ha reintrodotto nella società delinquenti non adeguatamente recuperati, ha determinato nuove situazioni di disagio per i cittadini e nuove sacche di delinquenza, aggravando ulteriormente le condizioni di sicurezza dei nostri territori. Finché la Lega farà parte integrante di questo Governo, non vi saranno indulti-manifesto o, peggio ancora, indulti mascherati. Siamo convinti che il problema delle carceri vada affrontato con lo spirito e con le iniziative messe in campo dal Ministro e dal Governo, ovvero attraverso un serio piano di edilizia carceraria di implementazione delle strutture esistenti, attraverso la costruzione di nuove carceri. Già all'epoca, negli anni 2000-2001, il ministro Castelli stanziò mille miliardi di vecchie lire per 1'edilizia carceraria

Sappiamo e abbiamo apprezzato il fatto che il ministro Alfano, insieme al ministro Maroni, in sede di Consiglio affari interni, abbia portato con determinazione e fermezza il problema delle carceri italiane, chiedendo un intervento immediato e risoluto delle istituzioni europee. I detenuti stranieri, gravano sullo Stato italiano per tre tipologie di costo: quello relativo alla sicurezza, quello economico per la celebrazione del processo

In conclusione, la Lega Nord è pronta a raccogliere tutte le sfide in tema di giustizia: non solo quelle relative alle carceri, dove sosterremo lealmente e con spirito di responsabilità le scelte del Governo mirate sicuramente a ridare dignità all'individuo, però all'insegna della certezza della pena, ma anche la sfida di una riforma organica, che tenga in seria e debita considerazione anche le vittime dei reati. Purtroppo tanto spesso, troppo spesso, ci ricordiamo e prestiamo attenzione a Caino dimenticandoci di Abele, perché esiste anche Abele. È spesso troppo semplice andare a visitare i carcerati, magari d'estate, come fanno alcuni colleghi dell'opposizione. Ricordiamoci invece di andare a visitare anche i cimiteri. Pensiamo a tutte le vittime spesso dimenticate, ai morti per mafia, per terrorismo, per rapina, ai morti per guida in stato di ebbrezza. dobbiamo pensare anche a quante vittime ci sono nel nostro Paese, a quanti famigliari di queste vittime stanno soffrendo, hanno sofferto e continueranno a soffrire per colpa di chi oggi è in carcere. Al tal riguardo, ricordo che da diversi mesi è depositato un disegno di legge a firma di tutti i senatori della Lega Nord, il n. 2590, per l'istituzione di un fondo di solidarietà a favore delle vittime dei crimini violenti. Signor Ministro, c'è tanto lavoro da fare. Auguri di buon lavoro da parte del Gruppo Lega Nord.

Signor Presidente, signor Ministro, qualche tempo fa una persona che lei conosce benissimo, il presidente del Consiglio ebbe a dire queste testuali parole: «La situazione nelle carceri è diventata intollerabile. Uno Stato civile non può togliere la dignità dalle persone. In passato il problema del sovraffollamento veniva risolto con amnistie e condoni, noi invece vogliamo dare una soluzione duratura nel tempo. Per la prima volta abbiamo deciso di dar vita a un piano per affrontare questa emergenza nelle carceri italiane. Ieri notte hanno dormito nei nostri istituti di detenzione più di 60.000 persone: la situazione è intollerabile». Questo diceva il *premier* Silvio Berlusconi annunciando il piano di emergenza sulle carceri approvato dal Consiglio dei ministri il 13 gennaio 2010. Oggi, a distanza di oltre un anno e mezzo, signor Ministro, lei ci è venuto nuovamente a raccontare di questo piano straordinario delle carceri per risolvere il problema del sovraffollamento nei nostri istituti penitenziari. Dunque, signor Ministro, anche se da poco si è insediato nel suo ruolo, è chiaro che non può non prendere coscienza che il piano carceri del suo predecessore e del premier Berlusconi è assolutamente fallito, è rimasto lettera morta. L'unica cosa che abbiamo di questo piano carceri di oltre un anno e mezzo fa è il sito «www.pianocarceri.it»: luogo virtuale nel quale i cittadini dovrebbero essere messi a conoscenza dell'avanzamento dello stato dei lavori degli istituti penitenziari. Peccato che questo sito sia la prova provata che il piano carceri del Governo Berlusconi è stato l'ennesimo *spot* elettorale, l'ennesimo *spot* di un Governo che dimostra di non avere alcuna attenzione nei confronti non solo della popolazione penitenziaria, ma neppure del personale che che lavora nei nostri istituti penitenziari. Possiamo però vedere sul sito - lo ripeto - «www.pianocarceri.it» i consulenti che sono stati incaricati dal precedente Ministro per studiare e poi realizzare

riferimento a intese, a decreti stralcio, ad accordi con le Regioni, ma nella sostanza sapeva benissimo che parlava di nulla. Il problema principale delle nostre carceri - come è stato già detto - è sicuramente quello del sovraffollamento. La popolazione penitenziaria è aumentata del 50 per cento negli ultimi tre anni e quindi è stato notevolmente superato il limite considerato regolamentare. È chiaro che, se aumentano i detenuti, ammesso che ci stiano fisicamente nei nostri istituti penitenziari, dovrebbe è banale, ma lo dico - aumentare anche il personale che in qualche modo deve occuparsi delle persone in carcere. Ma - come è già stato affermato in molti altri interventi il personale della Polizia penitenziaria è assolutamente sotto organico, e soprattutto è sottopagato. Sono di qualche mese fa alcune sentenze del TAR che hanno riconosciuto come dovuto giustamente il pagamento di ore di lavoro straordinario ad alcuni agenti della Polizia penitenziaria. Ma ancora più grave, se è possibile, è quanto viene detto di noi dalla Corte europea per i diritti umani. Sappiamo tutti che la Corte europea afferma che si è in presenza di tortura quando un detenuto è sottoposto a ristrettezza di spazi, ad assenza di luce, a privazione della libertà di lavarsi, all'esiguità delle ore d'aria, e purtroppo molti di questi fattori sono riscontrabili in diversi nostri istituti

più di 9.000 posti di nuova creazione ed una spesa di 600 milioni di euro, di cui non si è visto assolutamente niente. Signor Ministro, sicuramente la sua onestà intellettuale avrebbe dovuto portarla oggi a dirci qualcosa di più e di diverso da quanto il suo collega Alfano ha avuto modo di dirci oltre un anno e mezzo fa. I cittadini chiedono maggiore sicurezza e la politica spesso risponde con provvedimenti che sicuramente non sono adeguati e che spostano l'accento più sull'aspetto punitivo anziché su quello sociale di prevenzione e soprattutto pregiudicano fortemente la funzione riabilitativa

senza dimora e sofferenti psichici. Il carcere, dunque, come luogo di mera espiazione per chi è portatore di un disagio sociale, anziché luogo anche di rieducazione anche di rieducazione per chi ha commesso un reato come vorrebbe la nostra Costituzione. In dieci anni sono morte in carcere tantissime persone, oltre un terzo per suicidio e molte per cause ancora da accertare e che possono ricomprendere varie motivazioni: mancanza di assistenza sanitaria, *overdose*, incidenti di vario genere. Oggi per le persone recluse la speranza di uscire definitivamente da un circuito detentivo e quindi di effettuare un percorso di recupero si assottiglia sempre di più, perché mancano politiche che le incentivino e le sostengano nella ricostruzione della propria vita dopo la pena. Davanti all'abbandono e all'indifferenza sempre più spesso ci sono persone che non vedono altra possibilità che farla finita: quindi, signor Ministro, un fallimento per il nostro sistema carcerario che la nostra Costituzione individua come strumento reintegrativo dell'individuo all'interno della società. Nel nostro Paese ci sono emergenze che sicuramente meritano la prima pagina dei giornali: abbiamo visto questa estate l'emergenza rifiuti sulle strade di Napoli, barconi che scaricavano un'umanità variegata a Lampedusa, gli scontri in Val di Susa sulla TAV; però è stato importante che questa estate anche il fenomeno del sovraffollamento delle carceri sia stato portato all'attenzione dei cittadini e che i *massmedia*, anche se in

dobbiamo assolutamente sensibilizzare sempre di più l'opinione pubblica su questa emergenza. Sembra un'impresa colossale ma non lo è, e lo dobbiamo fare tutti insieme. tema di emergenza carceraria, anche negli interventi di questa mattina si è parlato di amnistia. È stato ricordato dalla Lega Nord anche l'indulto di qualche anno fa. Voglio ricordare ai colleghi senatori della Lega Nord che non solo loro votarono contro l'indulto, ma anche l'Italia dei Valori diede un giudizio negativo e un voto contrario a quel provvedimento. Parlando ora di amnistia, questa misura non appare convincente per varie ragioni, non ultima il fatto di essere una tipica misura emergenziale e quindi inidonea a risolvere strutturalmente il problema.

eludere una sentenza di condanna. Non credo quindi che l'amnistia, e tanto meno l'indulto, possano essere provvedimenti capaci di risolvere in modo organico il problema del sovraffollamento nelle nostre carceri. Vado a concludere, signor Ministro, con una preghiera. È chiaro che bisogna pensare a misure che si occupino, occupino, non a *spot*, ma in modo organico, della risoluzione della detenzione nelle carceri italiane.

riferiamoci agli ultimi anni - ha assunto, relativamente ai temi e alle problematiche dell'amministrazione della giustizia, un atteggiamento che è assolutamente distorto. È infatti chiaro che non si può pensare di risolvere il problema del sovraffollamento negli istituti penitenziari se non pensiamo anche ad altre misure che prevedano una riforma organica dell'amministrazione della giustizia. Uno Stato che intenda perseguire una repressione efficace dei delitti dovrà certo dotarsi di istituti penitenziari adeguati sia nel numero, sia dal punto di vista anche della qualità di vita, perché - ricordiamolo - la detenzione deve essere comunque accompagnata da un percorso di recupero del detenuto; ma anche del detenuto; ma anche i temi della giustizia, nel loro complesso, hanno necessità di una rivisitazione di tipo complessivo. Purtroppo, il Governo Berlusconi - non ce lo possiamo nascondere - non fa che parlare di processo lungo e prescrizioni brevi, ma non è mai in grado, come si suol dire, di prendere il toro per le corna. Esso, quindi, lascia senza risposte non solo i gravi problemi della giustizia, ma - innanzitutto - il problema delle carceri. Signor Presidente, intervengo alla luce di un dibattito molto intenso che si è svolto in quest'Aula su un tema particolarmente complesso e delicato, qual è - appunto - la condizione carceraria. Ritengo che sia giusto rimeritare i colleghi del Partito Radicale e Marco Pannella per questa iniziativa che - comunque - non può non trovare un Parlamento sensibile ai rilievi e, soprattutto, alla posizione che nel nostro ordinamento riviste la persona umana, sia essa anche condannata per un illecito penale. Si è discuto sulla funzione

importanti contributi che sono venuti dalla scienza criminalistica italiana, come quello di Cesare Beccaria, ma anche dalla scienza penalistica di altri Paesi, come per esempio il *probation* o il *parole*. In sostanza, questi interventi sui trattamenti penitenziari concernono sempre e particolarmente, non solo la rieducazione dei condannati, ma soprattutto la reintroduzione nel corpo sociale. Ho chiesto quindi la parola, signor Presidente, onorevoli colleghi, signor Ministro, soprattutto perché credo che, in prima analisi, occorrerebbe evitare - o comunque limitare - la fonte che genera una detenzione e una carcerazione così copiosa. penso che si possa ancora ragionare, nei termini di questa legislatura, su dei provvedimenti di modifica del codice penale, o comunque su interventi di depenalizzazione. Tuttavia, credo che non possa sfuggire a nessuno il rilievo in forza del quale il diritto alla sicurezza dei cittadini (quindi il diritto alla protezione contro la criminalità) sia un diritto parimenti importante, come pure il trattamento dei detenuti e dei carcerati. Ho chiesto, signor Presidente, onorevoli colleghi, signor Ministro, la parola perché non solo nella mia funzione di parlamentare, ma anche e soprattutto in quella di sindaco, sarebbe opportuno che nel trattamento dei detenuti si potesse avviare un percorso di coordinamento delle politiche assistenziali e di istruzione dei detenuti anche e soprattutto con le altre istituzioni che formano la Repubblica, quali appunto la Regione e, in particolare, i Comuni, a cui la nostra Costituzione attribuisce il servizio dell'assistenza. Credo quindi che se davvero vogliamo introdurre degli elementi di novità su questo dibattito, tenendo conto che la maggior parte dei nostri detenuti sono persone recidive e quindi il lavoro che occorrerebbe fare è appunto l'attività per prevenire le recidive, in particolare di reati molto gravi, tutto questo si possa fare coordinando le politiche di assistenza e di istruzione dei detenuti e dei carcerati, non solo prima che il reato sia commesso, quindi con funzione preventiva della criminalità, quanto e soprattutto a seguito della liberazione, spesso anche con misure clemenziali, come quelle che noi abbiamo vissuto e comunque che abbiamo conosciuto negli ultimi anni. Ritengo quindi, signor Ministro e onorevoli colleghi, che se da questo dibattito debba scaturire un provvedimento legislativo, questo debba essere coordinato nella Conferenza Stato-Regioni o Stato-Città per verificare nel concreto quali misure si possano apprestare per garantire a chi ha scontato una pena e deve essere ricondotto nell'ambito del consorzio sociale tutte quelle provvidenze e tutte quelle misure che siano capaci davvero di prevenire la ricaduta nel reato e quindi le recidive. Concludo, signor Presidente, onorevoli colleghi, dicendo che, nonostante quel che si è affermato in quest'Aula circa la presunta criminogenità

la criminalità ha ricevuto una sonora contrapposizione da parte delle forze dello Stato e della giustizia e oggi possiamo vantare il fatto che nel nostro Paese vi è un maggior livello di sicurezza e un minor numero di reati denunciati. *(Applausi del

ho sottoscritto subito e con convinzione la richiesta di convocazione straordinaria del Senato della Repubblica che i colleghi senatori Bonino, Perduca e Poretti hanno promosso secondo la procedura dell'articolo 62 della Costituzione. Ho ritenuto che, seppure in un tempo nel quale la politica non riesce più ad esprimere con compiutezza ed autorevolezza quella capacità di analisi e di guida che rispecchia la sua funzione primigenia, fosse tuttavia opportuno e giusto che il Parlamento svolgesse - per iniziativa dei senatori - una riflessione e che si confrontasse con il Governo su un tema così rilevante, quale quello della riforma strutturale della giustizia e dei rimedi da porre alla gravissima situazione in cui versa il sistema carcerario del nostro Paese. Certo, fino ad oggi in questa legislatura, i problemi della giustizia hanno occupato l'attenzione del Governo più per ritagliare strumenti legislativi estremamente parcellizzati e tesi a tutelare posizioni individuali (la prescrizione breve o il processo lungo: aggettivazioni antitetiche a seconda della necessità contingente) che per dare risposte ad esigenze collettive attraverso, appunto, riforme strutturali. In questi giorni, susseguendosi iniziative a livello nazionale e sui territori, l'attenzione si è fortemente catalizzata su questi argomenti, grazie anche - dobbiamo dirlo alla testimonianza di una personalità come Marco Pannella, coerente, anzi incrollabile interprete di una battaglia di civiltà che ha caratterizzato un lungo arco temporale del suo impegno civile, oltre che politico. Come pure va sottolineata la mobilitazione di associazioni e movimenti che hanno aderito da subito all'iniziativa dei radicali. Mi sono venuti in mente tre richiami forti che citerò in ordine cronologico: il primo data 23 marzo 1982, e cioè quasi trent'anni or sono,

Nell'Aula del Senato della Repubblica il senatore a vita Eduardo De Filippo pronuncia un memorabile intervento sulla condizione dei ragazzi dell'Istituto di osservazione per i minorenni «Gaetano Filangieri» di Napoli. Eduardo era impegnato - e tentò di coinvolgere anche questo ramo del Parlamento - a conseguire un obiettivo: l'integrazione nel tessuto sociale dei giovani dopo il periodo di istituzionalizzazione, «recuperando» - sono sue parole - «la speranza e la fiducia di una vita nuova che restituisca loro quella dignità cui hanno diritto e che giustamente reclamano».

abbia parlato nell'Aula di Montecitorio dinanzi alle Camere riunite in seduta congiunta, egli formulò una richiesta con riferimento alla situazione delle carceri nelle quali, cito testualmente, «i detenuti vivono spesso in condizioni di penoso sovraffollamento. Un segno di clemenza verso di loro mediante una riduzione della pena» - è sempre Giovanni Paolo II che parla - «costituirebbe una chiara manifestazione di sensibilità, che non mancherebbe di stimolarne l'impegno di personale recupero in vista di un positivo reinserimento nella società». Il 28 luglio di quest'anno - questo il presidente della Repubblica Giorgio Napolitano, intervenendo al convegno in Senato, più volte richiamato nel dibattito odierno, ebbe a dire: «È fondamentalmente dalla politica che debbono venire le risposte, (...) non escludendo pregiudizialmente nessuna ipotesi che possa rendersi necessaria». A mio avviso e secondo un'opinione diffusa, emersa a più riprese dal dibattito odierno, a parte i provvedimenti di amnistia e/o di indulto, che sono provvedimenti tampone che intervengono, per così dire, a valle del problema, occorre dar luogo ad interventi strutturali sulle pene e sull'esecuzione delle stesse. La politica della decarcerizzazione, assegnando alle misure restrittive in carcere una funzione residuale, deve prevedere oltre ad una ragionevole ed opportuna depenalizzazione, un sistema più articolato di sanzioni alternative, abbandonando il mito della "onnipotenza"

Naturalmente ciò richiede un congruo investimento sui servizi di sostegno ed una rete di solidarietà sociale idonea a sostenere i percorsi di *probation*: rapporti con il mondo dell'artigianato e dell'impresa per l'apprendistato, servizi dell'Amministrazione della giustizia integrati dai servizi territoriali degli enti locali, e così via. Cito Cito solo per titolo un altro tra gli innumerevoli problemi relativi alla condizione carceraria: la detenzione delle mamme e le delicatissime questioni connesse al loro rapporto con i figli durante il periodo di restrizione della libertà personale, nonché la necessità di rafforzare la rete di servizi integrati con l'apporto dei più appropriati specialismi, finalizzati ad alleggerire il trauma nei bambini e gli esiti devastanti che ne conseguono. Ho voluto soffermarmi più o meno esplicitamente soltanto su qualche aspetto dell'enorme problema che abbiamo innanzi. Intendo, in conclusione, evidenziare come e quanto a proposito della decarcerizzazione le misure alternative al carcere rispetto a determinati reati possano immediatamente offrire un primo rilevante rimedio al problema del sovraffollamento, così cambiando radicalmente l'approccio con il tema della detenzione: non più carceri, signor Ministro, trasformate in depositi sociali, usate come strumento per l'ordine pubblico. Di qui l'esigenza di un attento esame che porti alla depenalizzazione di alcuni reati. Una risposta, dunque, articolata, capace di incidere profondamente, e una volta per tutte su una problematica che interpella le nostre coscienze con quella prepotente urgenza richiamata dal Presidente della Repubblica, ma anche con una responsabilità che la politica, riappropriandosi del suo ruolo, deve assumere su di sé.

volevo osservare che questo dibattito, di straordinaria attualità e molto coinvolgente, almeno per quanto mi riguarda, e sono sicuro anche per gli altri, si è svolto su iniziativa di un gran numero di senatori, abbiamo una presenza ridotta a ranghi minimi. Il Ministro e i suoi Sottosegretari hanno diligentemente e con capacità di ascolto seguito tutti i lavori dall'inizio, così come diversi di noi, e parlo con non altro titolo se non quello di aver ascoltato diligentemente, data la materia, tutti gli interventi, ripromettendomi di ascoltare quelli che di certo mi seguiranno. Debbo anche anche osservare che sicuramente, per legittime esigenze dei colleghi e dei Gruppi, diversi di noi hanno visto anteporre numerosi oratori a quello che era l'originario schema al quale si erano rapportati. Aggiungo che diversi degli onorevoli colleghi, che hanno detto fra l'altro cose per me assai interessanti, dopo avere pronunciato il loro intervento hanno abbandonato l'Aula e se ne sono andati. se non vogliamo fare della demagogia spicciola (io non la faccio mai), è abbastanza comune ai lavori quando non si deve andare ad un voto, e non me ne faccio scandalo. in un'occasione come questa, se mi permette, signora Presidente (e sono certo di incontrare la sua personale sensibilità, non foss'altro perché è stata la prima promotrice dell'iniziativa), la questione non funziona così. Anche perché quando ben 140 e più senatori chiedono una seduta, i senatori debbo ritenere e presumere abbiano interesse ad ascoltare, voto o non voto, questo dibattito dal principio alla fine. Mi permetto allora di concludere, dopo questa considerazione agrodolce, che affido alla sua valutazione e a quella dei colleghi. quella dei colleghi. Coloro che per loro esigenze vogliano prendere la parola in questa seduta ovviamente non potranno che farlo, dato che sono le ore 18,10 e quindi siamo in pieno orario di lavoro; che coloro, come ad esempio il modestissimo sottoscritto, e sono certo altri qui presenti, preferiscano prendere dignitosamente la parola, per dignità

i colleghi siano a passeggio; credo e confido che, non solo Radio Radicale ovviamente, ma i sistemi di comunicazione interna possano consentire di raggiungere anche i colleghi Per quanto riguarda l'ordine dei lavori, la Conferenza dei Capigruppo, che ha definito le modalità di questa seduta, ha stabilito la continuazione del dibattito fino alle ore 20 e

attiene al tema se perdere il diritto alla libertà significhi oggi in Italia perdere, di fatto, tutti i diritti. Non essere più cittadini. Non essere, sostanzialmente, più umani. Come in molti hanno già detto, si può pensare di rimanere umani restando chiusi 22 ore su 24 in sette metri quadrati condivisi tra tre o spesso quattro persone? Si può dormire su strati di gomma che conservano nella forma, nel colore, nell'odore, l'impronta lasciata da migliaia di altri corpi nel corso di decenni? Si possono conservare la frutta, i biscotti, le altre derrate del cosiddetto vitto personale di fianco ai wc o fare la doccia (una volta ogni due settimane, anche d'estate) sotto un tetto di muschio, che pare quello di una caverna? descrivo una situazione precisa, quella del carcere della mia città, quella del carcere di Bologna. Ed è ponendoci queste domande che, con grave senso di frustrazione da impotenza per l'assoluta immobilità della situazione, (peggio, per la sua ingravescenza) insieme ad altre colleghe nel luglio scorso abbiamo chiesto la visita al carcere di Bologna della Commissione straordinaria per i diritti umani, costituita presso il Senato. Abbiamo in quell'occasione scattato l'ennesima fotografia di un incubo: 1120 persone (ordinariamente, in realtà, oltre 1200, perché il giorno prima della nostra visita era intervenuto uno "sfollamento" per per 70 detenuti), in un luogo progettato per 483, a cui è assegnata una capienza "tollerabile" (per chi, mi chiedo, tollerabile? In funzione di quale cambiamento sostenere tale tolleranza?) per 882 persone. Con loro vivono, di fatto "detenuti" anch'essi, 372 agenti di polizia penitenziaria, contro i 567 previsti dall' organico. Lei, signor Ministro, ha detto oggi che la capienza tollerabile complessiva degli istituti di pena in Italia esubera la popolazione carceraria, cioè che, sostanzialmente, i nostri istituti possono contenere tutti coloro che vi sono detenuti e che avanza perfino qualche spazio. Ma non è sulle valutazioni medie o sulle valutazioni complessive che si può misurare l'umanità o la sostenibilità di una condizione. È sulla condizione soggettiva in cui ciascuno vive. Anche in occasione della visita della Commissione diritti umani abbiamo faticato a rintracciare il senso della nostra azione, così come ogni volta in cui abbiamo interrogato il Governo (sette volte negli ultimi tre anni), senza mai ricevere risposta. Abbiamo ritenuto comunque che un filo di senso potesse essere ritrovato nel mantenere accesa una luce, nel mantenere viva l'idea che il carcere è a pieno titolo una comunità parte di un'altra comunità, la città. Perché questo non rimanga una mera affermazione di principio tanto facilmente condivisibile, come abbiamo visto qui oggi, quanto sterile, occorre che almeno alcuni interventi di cambiamento minimo siano attuati immediatamente al termine di questa sessione dei lavori e che prima di ogni grande riforma, di cui da tanto si parla, ma che mai è stata affrontata, siano almeno realizzate alcune precondizioni di civiltà. Innanzitutto, a proposito della dimensione civica delle carceri, è irragionevole ed immotivato che ai sindaci, massima autorità sanitaria delle città, non sia riconosciuto il medesimo diritto di accesso e funzione ispettiva presso le carceri che è riconosciuto ai parlamentari e ai consiglieri regionali; ciò in ragione non solo del pieno esercizio della funzione di garanzia sulle condizioni di salubrità della comunità carceraria, ma per mantenere vivo, simbolicamente e fattualmente, un rapporto di integrazione del carcere con la città, che è alla base dell'attuazione di progetti fondamentali per realizzare la funzione educativa della pena. C'è una proposta di legge, depositata in Parlamento, che va in questo senso; non costa nulla: approviamola subito. Così come è utile approvare, finalmente, la legge istitutiva del Garante nazionale dei diritti delle persone private della libertà: i numerosi progetti depositati e discussi non richiedono che una decisione finale, che siamo in grado di prendere e che sarebbe di buon supporto a quelle autonomamente prese in questo senso da molte municipalità. In secondo luogo è non solo inaccettabile ma sostanzialmente irragionevole che, a fronte di un incremento costante della popolazione penitenziaria, si siano agiti in un triennio tagli ai trasferimenti per il mantenimento degli istituti che ne rendono impossibile la conduzione anche in regime ordinario. Del tema delle risorse, signor Ministro, lei oggi non ha ritenuto di parlare. Pochi numeri (parlo sempre del carcere della mia città): il bilancio complessivo del carcere di Bologna in tre anni è stato decurtato del 55 per cento. Dal 2008 al 2011 sono stati tagliati del 25

L'11 luglio scorso la direttrice del carcere ci comunicava che erano rimasti in cassa 60.000 euro e che, da settembre, si sarebbe potuta verificare una difficoltà sostanziale a garantire il pagamento della fornitura delle derrate destinate alla realizzazione del vitto per i detenuti; due sole alternative possibili: affamarli o non pagare i fornitori, come già di fatto avviene ad esempio con le forniture della società municipale per l'erogazione del servizio idrico e delle Un altro dato drammatico riguarda il lavoro in carcere e dopo il carcere. La riduzione dei fondi ha determinato già nel 2010 il dimezzamento delle ore impegnate (da sei ore medie a 3 ore giornaliere) di ciascuno dei già pochissimi lavoranti: solo 100 detenuti su 1200, infatti, a Bologna sono impiegati in attività lavorative all'interno del carcere, peraltro indispensabili per il funzionamento dei servizi minimi: la produzione dei pasti, le pulizie, lo smaltimento dei rifiuti. I detenuti impegnati in attività formative non superano il 10 per cento. Quella della formazione e del lavoro è l'esigenza più sentita dai detenuti, come emerge chiaramente dal verbale di visita della Commissione diritti umani. Creare un modello carcerario in cui il lavoro rappresenti un fondamentale strumento di rieducazione delle persone sottoposte a pena detentiva, nel pieno rispetto di quanto previsto dall'articolo 27 della Costituzione, non sembra un obiettivo impossibile. Sono diverse le proposte depositate in Parlamento che portano firme di autorevoli autorevoli rappresentanti di tutti i Gruppi politici. Ne cito una, fra tante, a prima firma del senatore Treu e del presidente Gasparri. Occorrerebbe andare in questa direzione e trasformare i servizi minimi che i

La riduzione dei casi di recidiva comporta l'abbattimento dei costi sociali derivanti dalla commissione dei reati e dei costi economici legati al mantenimento delle carceri. Per ogni punto di abbattimento delle percentuali di recidiva si stima che lo Stato possa risparmiare fino a 60 milioni di euro l'anno per le sole spese di giustizia, per il minore utilizzo di forze dell'ordine, per minori spese di amministrazione penitenziaria, per le spese sanitarie. Un investimento in questa direzione è destinato, quindi, ad autosostenersi, sia in termini economici che in termini sociali. Infine, un'ultima considerazione relativa alla realizzazione del Piano carceri. Anche a Bologna è prevista la realizzazione di una nuova struttura detentiva per 200 posti. Ritengo però che la realizzazione di nuova capienza sia in contrasto sostanziale con la necessità di utilizzare la detenzione con criteri di assoluta appropriatezza, che sono perseguibili evitando la carcerazione dei sofferenti psichici e dei tossicodipendenti, limitando la legislazione crimonogena in materia di immigrazione, potenziando al massimo le misure alternative ed agendo, come descritto, verso la prevenzione. Mi limito in questa sede ad una considerazione di buon senso: non si può pensare di destinare nemmeno un euro alla realizzazione di nuovi muri per recludere prima di aver reso quelli esistenti salubri, sicuri, vivibili. Il dubbio che sorge è che le ingenti risorse destinate alle nuove realizzazioni (se mai si faranno) rinvengano, paradossalmente, dalla riduzione dei fondi destinati alla gestione alla gestione ordinaria. Vi chiediamo perciò - lo chiediamo a lei, signor Ministro - di riflettere seriamente su quale sia l'investimento più coerente in nome della sobrietà e della salvaguardia di una comune umanità.

L'ho apprezzato quando ha sottolineato il problema delle traduzioni, un problema grave che conosco bene perché prima gravava tutto sulle Forze dell'ordine, paralizzandole, e soprattutto quando ha indicato alcune soluzioni possibili per risolvere il dramma dei malati di mente reclusi in luoghi indegni di un Paese civile.

e che non lo considera un ostacolo al fare del Governo, come qualcuno ha detto qualche tempo fa. Ho inoltre apprezzato l'impegno assunto di realizzare nuovi posti, migliaia di posti, nel 2012. L'augurio che mi faccio e che rivolgo

rischio di essere ripetitivo, ma l'argomento è così importante che mi fa piacere anche essere ripetitivo. Le osservazioni critiche che sto per porre, onorevole Ministro, non riguardano la sua persona. Ha ragione il collega D'Ambrosio a dire che si aspettava proposte e soluzioni,

chi l'ha preceduto, che ha avuto costantemente inerzia nella sua attività, mirando soprattutto a certi obiettivi? Per inquadrare l'emergenza che grava sul nostro sistema carcerario basta ricordare ancora una volta (lo faccio ancora) i dati resi noti dall'amministrazione penitenziaria, diffusi dalla stampa e citati più volte da chi mi ha preceduto: quasi quasi 25.000 detenuti in più rispetto ai posti letto regolamentari. In una logica di confronto costruttivo, visto che lei ha proposto di lavorare insieme,

un individuo vive in meno di tre metri quadrati, laddove il Consiglio d'Europa ne prevede 4 nelle celle multiple e 7 singole,

quasi il 45 per cento della popolazione carceraria trattenuta in via cautelare, dunque senza aver ancora subito una condanna definitiva, un dato questo che non ha pari nell'Unione europea e che ci vede appaiati alla Turchia e a Cipro; 47 suicidi in carcere dall'inizio dell'anno, di cui due lo scorso fine settimana, e da ultimo la sentenza con cui il tribunale di sorveglianza ha condannato l'amministrazione penitenziaria del carcere di Borgo San Nicola a Lecce a risarcire un detenuto per l'insostenibile sovraffollamento degli spazi in cui vive. Un disastro. Un disastro senza dubbio annunciato, dal momento che la stessa situazione si è riproposta innumerevoli volte negli ultimi anni ed è stata sempre affrontata con provvedimenti emergenziali (l'indulto *in primis*), mai risolutivi. Il carcere in Italia, lungi dall'essere la palestra rieducativa che tutti dovremmo augurarci, come prevede la Costituzione, è luogo di mortificazione e vendetta, dove ogni differenza viene annullata senza logica né giustizia: autori di reati dolosi, colposi, delitti di sangue, reati contro il patrimonio, mafiosi, tutti costretti nelle medesime condizioni. Gli allarmi, anche in sedi autorevoli, si sono moltiplicati negli ultimi mesi; bene ha fatto lei a ricordare l'appello del Presidente della Repubblica, eppure il Governo ha fatto poco o niente su questo tema. Qui desidero rivolgere un saluto e un ringraziamento all'onorevole Pannella, a lei, presidente Bonino, e al Partito Radicale per aver fatto riemergere il problema dall'indifferenza istituzionale che lo avvolge. Le sporadiche iniziative che ha preso l'Esecutivo sono rimaste lettera morta. È questo il caso del piano di potenziamento dell'edilizia carceraria, del programma di adeguamento dell'organico della Polizia penitenziaria, entrambi in attesa di realizzazione. La mancanza di personale, proprio per l'*iter* burocratico che bisognava seguire, ha di molto ridotto anche l'impatto del cosiddetto svuota-carceri, l'unica misura legislativa seria adottata da chi l'ha preceduta. Il provvedimento, infatti, non ha risolto il problema e ha fatto sì che solo 2.400 persone lasciassero gli istituti. Da dove partire allora? Sicuramente da un sostanzioso investimento umano e finanziario che consenta la creazione di nuovi posti - lei lo ha lo ha sottolineato - mettendo innanzitutto in funzione strutture già esistenti (Pinerolo, Sassari, San Valentino in Abruzzo, Monopoli e altri) che ad oggi non è stato possibile aprire per mancanza di operatori specializzati e fondi. La gravissima crisi finanziaria non sfugge a nessuno, è nota a tutti, ma ci sono settori, come la giustizia e la sicurezza, sui quali in nessun frangente è possibile risparmiare. Allo stesso tempo, è indispensabile rivedere tutta la nostra politica criminale, lavorando a monte perché il numero dei detenuti non aumenti, anziché a valle quando il sovraffollamento delle carceri è divenuto insostenibile. Un'analisi dei tipi di reato che oggi si scontano nelle prigioni italiane potrebbe aiutare a muovere i primi passi in questa direzione. La maggioranza dei detenuti ha commesso reati contro il patrimonio o legati alle sostanze stupefacenti. Per entrambe le tipologie, dopo accurata selezione caso per caso, si possono applicare sanzioni alternative - lei lo ha previsto - alla detenzione, sanzioni di tipo amministrativo o, nel caso dei tossicodipendenti, percorsi di reinserimento sociale. Non dobbiamo temere la depenalizzazione di alcuni reati se le alternative sono ben impostate ed attuate. richiede poi la categoria dei detenuti immigrati che, in molti casi, affollano gli istituti di pena per qualche ora o per qualche giorno per non aver ottemperato all'obbligo di espulsione o di allontanamento. Signor Ministro, non si faccia anche lei prendere la mano da chi anche oggi ha ripetuto che l'immigrato è la causa di tutti i mali del nostro Paese. Guardi che cosa hanno combinato a Lampedusa

La loro breve permanenza carceraria manda il sistema in *tilt* - lei, da magistrato, prima ancora che da Ministro, sa bene cosa sto dicendo - senza alcuna utilità. Una stortura che è in gran parte dovuta alle norme sull'immigrazione, varate con gran clamore mediatico da un Governo più interessato a mantenere il consenso di una parte dei suoi elettori che non a risolvere i problemi del Paese.

Si tratterebbe di un'autorità indipendente, di un garante nazionale la cui istituzione è stata richiesta e sollecitata dalle Nazioni Unite attraverso il Protocollo alla Convenzione contro la tortura, che l'Italia ha firmato nel 2003 e non ha mai ratificato, proprio perché entro un anno si sarebbe dovuta dotare di tale autorità. Il monitoraggio continuo ed ufficiale degli istituti di pena è infatti premessa indispensabile per il funzionamento del sistema penitenziario. Non è ammissibile che il luogo di esecuzione delle pene, quindi dell'applicazione della legge, sia esso stesso al di fuori della legalità, rendendo la funzione rieducativa della pena pura utopia. Sotto il profilo normativo è inoltre indispensabile introdurre il delitto di tortura nel codice penale. La relativa convenzione risale al 1984; l'Italia l'ha ratificata nel 1987 e, nonostante i numerosi tentativi, non l'ha ancora messa in atto. Cari colleghi, onorevole Ministro, resta infine il fatto che nessun cambiamento incisivo in tema di politica carceraria è possibile se contemporaneamente non si procede a una riforma globale della giustizia. Chi più di lei, Ministro, sa questo? Il cambio di guardia al Ministero ci lascia in tal senso ben sperare. predecessore, che aveva come unico obiettivo la salvaguardia degli interessi giudiziari di qualcuno, ha generato mostri. La parte politica che rappresento ha tentato di inserire nella manovra finanziaria appena varata un pacchetto sulla giustizia che muoveva i primi passi di una riforma sempre annunciata e mai neanche pensata. Abbiamo proposto la revisione delle circoscrizioni giudiziarie, secondo il criterio di un tribunale per ogni provincia, il sostegno all'informatizzazione (ancora a zero, a dispetto delle affermazioni fantasiose di qualche Ministro), con particolare riguardo alla promozione dell'uso della posta certificata per le notifiche, sia civili che penali. E, soprattutto, abbiamo presentato un emendamento sulla modifica dell'articolo 81-*bis*, finalizzato ad accelerare i tempi del processo civile e a sanzionare i comportamenti dilatori di avvocati, giudici e consulenti. Solo quest'ultima proposta, anche grazie al suo intervento, Ministro, è stata accolta, mentre sul resto abbiamo trovato un muro. Non è a lei, onorevole Ministro, che devo spiegare in che condizioni versano i tribunali italiani, sommersi di carte, persi in calendari infiniti che rendono il processo civile interminabile e violano il principio costituzionale del giusto processo. Le lungaggini giudiziarie sono una zavorra per la crescita del Paese e lo stesso Governatore della Banca d'Italia, nella sua ultima relazione, individua la riforma della giustizia e dei tempi della stessa come un'assoluta priorità per la crescita dell'Italia.

è vero che dopo tanti interventi potrei rischiare di essere ripetitiva, ma l'argomento è tale che va onorato dibattendo, anche contando sul fatto che molti dei nostri colleghi siano nei propri uffici ad ascoltarci.

quella di essere occasione di recupero sociale e di riscatto individuale. Certamente è necessario governare il problema - come è stato autorevolmente detto

In certe situazioni, descritte anche durante questo dibattito dai colleghi che mi hanno preceduto, il recupero è spesso impossibile.

dove solo la grande professionalità degli uomini della Polizia penitenziaria, il loro spirito di sacrificio e abnegazione malgrado organici sottodimensionati - questo è un grosso problema

La certezza della pena, dunque, ma anche la sua efficacia per il recupero della persona, va garantita attraverso una condivisione di vita che non sia quella che attualmente si riscontra nelle prigioni. Tuttavia penso che ai problemi delle carceri non si debba rispondere con amnistie, indulti o depenalizzando reati come lo spaccio di droga. Solo la presente la presente emergenza può giustificare, e semmai far accettare, la richiesta avanzata dalla presidente Bonino nel suo intervento introduttivo. Infatti, la fallimentare esperienza dell'indulto del Governo Prodi ne è l'ultima esemplare conferma: dopo pochi mesi molti dei detenuti liberati sono di nuovo tornati nelle carceri. Per evitare il sovraffollamento, si richiede la messa in campo di un ventaglio articolato di misure, a partire, certamente, dalla predisposizione di nuove strutture carcerarie dall'assunzione di altri agenti di custodia, da un'intelligente depenalizzazione e da un ricorso alla carcerazione preventiva solo nei rigorosi nei rigorosi limiti fissati dalle norme. Nell'immediato, sarebbe però auspicabile tentare di far diminuire la popolazione carceraria piuttosto che chiedere forti investimenti, che non sempre sono disponibili, in nuove carceri, anche se indispensabili, che hanno certamente tempi di lunga realizzazione. È allora indispensabile potenziare l'azione di prevenzione delle forze dell'ordine. La prevenzione, sulla quale dobbiamo lavorare e che ha un costo, è un onere sociale ed economico sicuramente inferiore a quello della punizione. Di un caso occorre parlare: quello delle tante persone in attesa di giudizio, detenute a volte per anni. Eliminare questa situazione, fondamentalmente ingiusta, farà diminuire la popolazione carceraria. Ciò sarà possibile, all'interno della riforma della giustizia, attivando strumenti processuali che evitino lunghe permanenze in prigione. Occorre anche operare per evitare l'attuale uso diffuso delle carcerazioni preventive, utili solo a tenere a bagnomaria persone non colpevoli fino a prova contraria, per indurle a soddisfare le necessità degli inquirenti, spesso ispirate - purtroppo lo abbiamo visto molte volte - a pulsioni mediatiche. Come ho detto, ritengo ingiusto depenalizzare reati come lo spaccio di droga. Sarebbe invece giusto trovare alternative sicure e che offrano occasioni di recupero ai tossicodipendenti che spacciano. Costoro, da soli, rappresentano una buona parte dell'attuale affollamento carcerario, signor Ministro. Per ottenere questo risultato, sarebbe necessaria la massima collaborazione tra le strutture dello Stato. Al contrario, accade che una Regione paghi la retta ad un centro di disintossicazione e recupero, dove potrebbero essere inviati i tossicodipendenti spacciatori, solo per i residenti della Regione È quanto avviene nella mia Umbria, dove la Regione dà ai centri di recupero e di prevenzione rimborsi solo per i residenti nella Regione. Credo che si potrebbe attivare lo stesso sistema usato per la migrazione sanitaria, cioè le Regioni anticipano la spesa salvo compensare i costi con l'ente della Regione di provenienza. Questo potrebbe farsi, signor Ministro, perché c'è un certo disagio all'interno dei centri di recupero. L'affollamento delle carceri diminuirà oltremodo mettendo in atto un'azione di vasto respiro da parte di tutte le agenzie educative, per dare ai giovani quei valori che sono il primo scudo protettivo contro i comportamenti antisociali. Una valutazione, infine, vorrei fare per i detenuti stranieri, sui quali molti si sono intrattenuti, che rappresentano - ci ha detto il Ministro - il 36 per cento dell'attuale affollamento carcerario. Penso che per costoro la misura più efficace sia il rimpatrio immediato, tra l'altro a costi certamente inferiori rispetto alla permanenza nelle nostre carceri. Ci sono già leggi e misure in questo senso che, a mio avviso, vengono eluse o poco utilizzate. La prigione - concludendo - dovrebbe essere l'ultima spiaggia per chi ha deviato dalla correttezza sociale. Essa deve tornare ad essere luogo di recupero e reinserimento dove chi entra delinquente ne possa uscire riabilitato alla vita sociale.

Signora Presidente, queste sono giornate molto difficili per l'Italia, che improvvisamente si è scoperta con una pessima reputazione sia per quanto riguarda i rischi di solvibilità del suo debito che per l'affidabilità dei suoi governanti. Ciò nonostante, ho voluto sostenere - l'ho fatto con convinzione - l'iniziativa della vice presidente Bonino per la convocazione straordinaria di questa sessione dell'Aula. Penso infatti che parlare di carcere e di giustizia non sia parlare d'altro rispetto alla crisi italiana e che riformare la giustizia e aggredire la drammatica situazione di sovraffollamento delle carceri italiane significhi anche operare per il risanamento dei conti pubblici e favorire la crescita del sistema Italia. Esistono peraltro studi economici e simulazioni contabili in questo senso. L'ultima che ho potuto vedere sostiene la superiorità degli strumenti fiscali nel contenere il consumo di droghe rispetto all'applicazione di una normativa proibizionista e penalista. In Italia il consumo di tabacchi e di alcolici è per l'appunto scoraggiato da un'elevata tassazione. Se anche il mercato delle droghe fosse trattato come quello dei tabacchi avremmo certamente un forte beneficio fiscale. Avremmo un risparmio di circa 2 miliardi l'anno per le spese, tanto costa l'applicazione della normativa proibizionista in merito a Polizia, magistratura e carceri, e con un ricavo derivante dalle imposte sulla vendita della sola *cannabis* di circa 5 miliardi e mezzo l'anno. Tutto ciò senza considerare i vantaggi di legalità e crescita economica che questa porterebbe con sé. Purtroppo però è proprio questa visione delle riforme che sarebbero necessarie che Governo e maggioranza hanno dimostrato di non avere e di non riuscire a perseguire. È per questo che ieri, visitando il carcere di Poggioreale e parlando con molte persone detenute, che nutrivano grandi aspettative da questo dibattito parlamentare, ho sentito la responsabilità ed il dovere di non alimentare troppo queste aspettative, senza tuttavia sottrarre speranza. Una speranza che vive nel nostro impegno parlamentare ma soprattutto nella volontà decisionale del Governo, e che perciò è tutta da dimostrare anche nelle parole del Ministro che spero saranno più incisive nella parte conclusiva del nostro dibattito. Signor Presidente, le carceri sono un pezzo importante e integrante della vita della mia città. Napoli, come poche altre città, vive un'osmosi forte tra carcere e territorio e la vita nel carcere ci può dire molte cose della città stessa. La casa circondariale di Poggioreale vede un transito annuale di 15.000 ingressi, è una città nella città. Il problema più grave è quello del sovraffollamento che a Poggioreale significa 2.634 detenuti, a fronte di una capienza regolamentare di 1.400, due terzi in attesa di giudizio, un quarto (670) tossicodipendenti, 270 detenuti di alta sicurezza. Per quanto riguarda i detenuti stranieri, è stato interessante verificare che sono meno del 10 per cento, in distonia rispetto al dato nazionale. Altri problemi sono altrettanto gravi. Gli agenti di Polizia penitenziaria in servizio sono 730 (dovrebbero essere 950) e operano su 3 turni. La caserma per gli agenti versa in particolari condizioni di precarietà così come l'impiantistica di sicurezza. Ma soprattutto ciò che emerge sono le conseguenze gravissime del taglio delle risorse finanziarie che incide persino sulla manutenzione ordinaria di strutture peraltro vetuste e sugli approvvigionamenti di generi di prima necessità. La precedente Giunta regionale aveva finanziato un campo di calcetto, che è stato realizzato migliorando davvero di poco la carenza strutturale di spazi di socializzazione. Altri finanziamenti precedentemente stanziati sono i 600.000 euro finalizzati alla ristrutturazione di laboratori di falegnameria, tipografia e officina che sono stati però distolti dall'attuale governo regionale, con il risultato di deprimere ulteriormente la possibilità di lavorare per tanti detenuti. Dieci anni fa erano 400 i detenuti che lavoravano, oggi sono solo 140 e per tutti gli altri non ci sono possibilità di lavoro e di guadagno (naturalmente neanche fuori, siamo a Napoli), a Napoli), fattori importantissimi ai fini del recupero sociale in una città come la nostra. Anche per quanto riguarda il diritto alla salute dobbiamo dichiarare di essere fuori dalla Costituzione. Si sa che il diritto alla salute versa in condizioni critiche per tutti i cittadini napoletani, ma nel caso dei detenuti la negazione di questo diritto va denunciata con particolare vigore e le soluzioni devono essere oggetto di specifiche iniziative e percorsi garantiti. Infatti, mentre qualunque cittadino potrà recarsi in ospedale anche fuori Regione, se necessario, ai cittadini ristretti nella libertà di movimento lo Stato deve garantire l'accesso agli ospedali, e questo purtroppo oggi non avviene. Anche l'istituto penale per i minori di Nisida, ubicato in uno dei siti più suggestivi al mondo, che per questo potrebbe e dovrebbe essere destinato ad altro uso in una città tanto carente di spazi pubblici e risorse, vive gli stessi problemi. Al momento della mia visita erano presenti 50 ragazzi e 10 ragazze: la popolazione naturalmente era in soprannumero e - mi si è detto - quasi raddoppiata negli ultimi anni. La maggior parte dei minori detenuti è napoletana, ad eccezione - questo mi ha molto colpita - della componente femminile, composta esclusivamente da ragazze rom, con reati minori come furti di appartamento. Rom, immigrati e tossicodipendenti affollano i nostri istituti di pena e testimoniano, così come il penoso permanere degli OPG, la decadenza di civiltà giuridica e democratica del nostro Paese. Gli OPG rappresentano un vero e proprio oltraggio alla coscienza civile per le condizioni aberranti in cui versano 1.500 nostri concittadini, 350 dei quali dovrebbero già essere usciti. uno scandalo a cui il Governo deve porre fine immediatamente: per altro, può e deve farlo all'interno della normativa attuale. Signora Presidente, le nostre carceri stanno per scoppiare. In questo momento l'Italia, con la Bulgaria, ha le carceri più affollate d'Europa. Se applicassimo una misura alternativa almeno alla metà dei detenuti con un fine pena inferiore a tre anni, il numero dei detenuti scenderebbe a 55.000. Se poi decidessimo, fino in fondo, di praticare la via di misure alternative, anche sperimentali, potremmo spingerci oltre il carcere, a cominciare, per esempio, dal superamento dei penitenziari femminili. I dati ci dicono che le donne delinquono meno degli uomini: infatti, sono il 4 per cento del totale della popolazione carceraria, con reati prevalenti del tipo di violazione del patrimonio e droga. Si potrebbe spendere molto meno chiudendo costosissimi penitenziari e garantire molto meglio sia l'espiazione della pena, che il recupero attraverso altri percorsi. II sovraffollamento non c'è per caso, ma per causa di leggi che hanno un nome ed un cognome, come quelle sulle droghe, sull'immigrazione e sulla recidiva. Da sola, la legge sulle droghe riempie la metà delle carceri italiane. In Europa tutti - anche chi ha le leggi più punitive - sostengono che le persone tossicodipendenti non devono stare in carcere. Da noi, invece, accade il contrario. Misure alternative alla detenzione, semilibertà e lavoro esterno, piani di lavoro socialmente utili: questo è tutto quello che serve fare e, per farlo, è urgente un piano finanziario con risorse finalizzate, impegnando, ad esempio, quelle inutilmente congelate nella cassa delle ammende. Noi crediamo che tutto questo possa e debba essere fatto, così come misure di depenalizzazione, limitazione e riforma della custodia cautelare. Penso che sia giusto accompagnare questo programma con una misura vasta di amnistia, che rappresenti il completamento di una più ampia azione di riforma e non solo un provvedimento a se stante.

mi pare che ci sia ancora un *misunderstanding*. Ho apprezzato le parole del Ministro che convergono sul lavoro che ha fatto e che sta facendo la Commissione d'inchiesta. Io sono relatore del provvedimento sugli OPG insieme al senatore Saccomanno. Proprio

quello carcerario è uno degli aspetti che non è mai cambiato in Italia. Probabilmente, dalla proclamazione del Regno d'Italia ad oggi il sistema carcerario è rimasto per alcuni versi immutato; talvolta, anche le mura sono rimaste immutate.

legato al carcere. Sappiamo che, se si accentua l'aspetto punitivo e non quello rieducativo, se il detenuto non viene reintegrato dal punto di vista lavorativo durante la sua permanenza in carcere, quando uscirà c'è un costo sociale elevatissimo perché quel soggetto non si reintegra e ritorna a delinquere. C'è un costo elevatissimo di strutture socio-assistenziali a causa di un sistema carcerario, come quello di oggi, troppo punitivo. E poi vi è un costo economico. Un carcerato costa grosso modo come una giornata di riabilitazione sanitaria in una struttura ospedaliera. Mi pare un po' troppo, anche perché qui, purtroppo, non si riabilita proprio nulla. Da anni rincorriamo questa emergenza in due modi: o con le amnistie e gli indulti o con la costruzione di nuove carceri. C'è questa corrente alternata. Non riusciamo probabilmente a trovare una modalità corretta per regolarizzare un sistema. Ho apprezzato il fatto che si stanno spendendo 350 milioni di euro e che, a fine 2013, avremo nuove strutture pronte; apprezzo moltissimo il discorso delle strutture a bassa sicurezza, tra cui anche quella di Pavia, la città dove vivo. Peccato che il nuovo carcere, progettato per sfruttare al massimo gli spazi, utilizzerà gli spazi comuni del vecchio carcere, per cui si raddoppiano i detenuti ma gli spazi comuni rimangono gli stessi

Il Presidente della Repubblica, intervenendo nel convegno dal titolo «Giustizia! In nome della legge e del popolo sovrano», il 28 luglio scorso, ha delimitato a mio avviso anche il campo dell'attuale dibattito nel "mettere a fuoco il punto critico insostenibile cui è giunta la questione, sotto il profilo della giustizia ritardata e negata, o deviata da conflitti fatali fra politica magistratura, e sotto il profilo dei principi costituzionali e dei diritti umani negati per le persone ristrette in carcere, private della libertà per fini o precetti di sicurezza e di giustizia".

Ed è questa la linea che cercherò di seguire nel mio intervento. Parto dal primo punto: il presidente Napolitano ha dichiarato che riteneva già esaustivi gli interventi più volte espressi nel corso del mandato tesi ad esprimere preoccupazioni ed esigenze relative sia al superamento di gravi inadeguatezze e insufficienze del "sistema giustizia" in Italia sia al rispetto degli equilibri costituzionali nel rapporto tra politica e giustizia. Ebbene, Ministro, sono stati davvero ascoltati dal Governo questi appelli? Io credo di no, perché se così fosse non ci troveremmo nella situazione di dissesto della giustizia penale (tratterò oggi solo di questa) la cui (voluta) inefficienza si riflette anche sul pianeta carcere. Volutamente il tema della riforma della giustizia è stato posto in questa legislatura facendo confusione tra il piano dell'efficienza, dei tempi, della qualità della giustizia e quello del «riequilibrio» tra i poteri per ridimensionare la giurisdizione, giocando sull'ambiguità di sovrapporre due piani, che hanno ben pochi punti di contatto. In questo modo l'attenzione del Governo e della maggioranza ha potuto soffermarsi su ben altre priorità che efficienza e durata: inizialmente sulla legge cosiddetta bloccaprocessi del 2008, poi sulla tematica delle intercettazioni (non garantendo la *privacy*, depotenziando lo strumento investigativo e comprimendo la libertà di informazione). Ed è seguito, quindi, in un crescendo, il disegno di legge sulla riforma del processo penale, il disegno di legge n. 1440, con l'intento di incidere sui rapporti tra pubblico ministero e polizia giudiziaria, per culminare nel processo breve e oggi nella prescrizione brevissima per gli incensurati, accompagnata dal contemporaneo e contraddittorio disegno di legge (nato con altra finalità) di riconoscere all'imputato il diritto a far dilatare i tempi del processo in materia di prove per guadagnare la prescrizione (il cosiddetto processo lungo). Sorvolo sulla riforma costituzionale che, tesa a minare l'indipendenza e l'autonomia, si è giustamente impantanata alla Camera sul cosiddetto lodo Alfano, dichiarato incostituzionale con sentenza n. 262 del 2009, e sulla successiva legge sul "legittimo impedimento", (dichiarata parzialmente incostituzionale il 13 gennaio 2011 e poi, definitivamente, cancellata dal *referendum*). Sono così trascorsi, signor Ministro, tre anni di legislatura inutili senza che alcuna riforma strutturale, ordinamentale, penale, sostanziale e processuale sia stata posta in essere per rendere la giustizia efficiente e veloce e intervenire, in conseguenza, anche sulle distorsioni del sistema carcerario: senza porre in essere alcuna precondizione, come ha dichiarato giustamente oggi la senatrice Bonino, per poter prendere in considerazione l'opportunità di un provvedimento di amnistia come un rimedio a questo disastro. L'amara constatazione è che il dibattito su questi temi ha avuto solo l'effetto di sottrarre tempo al Parlamento e di distogliere l'attenzione dalla stringente necessità di interventi strutturali tesi a realizzare un processo uguale per tutti e in tempi ragionevoli e ad affrontare, contemporaneamente, in modo serio, organicamente, la drammatica situazione carceraria. Le chiedo allora, signor Ministro, di chiarirci in questa sede se intende avallare questa strategia di destrutturazione della giustizia o imboccare la via delle riforme strutturali per ridurre i tempi dei processi e incidere sulla realtà carceraria le dico che mi aspetto da lei questa seconda risposta). Se così è, Ministro, lei comunque nulla ci ha detto al riguardo. Anzi, è partito dalla volontà di evitare ogni contrapposizione, ogni polemica, per dirci che, sì, è vero, non vi devono essere cedimenti rispetto ai valori costituzionali, per cui nel carcere deve essere assicurato l'ordine, deve essere garantita la salute e imposto sotto il profilo logistico il sereno svolgimento dell'espiazione della pena o della custodia cautelare, ma, tutto sommato, malgrado uno scoperto di organico della Polizia penitenziaria di ben 5.877 unità (che non ci ha spiegato come intende sanare), malgrado la clamorosa carenza degli educatori (fatto su cui nulla ci ha riferito), e un bilancio della riforma della sanità che ha maggiore difficoltà di garanzia dei precedenti livelli di efficacia e continuità assistenziale medico-infermieristica nelle Regioni interessate ai piano di rientro debitorio, i 206 istituti penitenziari esistenti consentono una presenza regolamentare di 45.732 detenuti ed una tollerabile presenza di 69.164 detenuti, onde, essendone presenti 67.377, si è a circa 2.000 detenuti sotto la soglia di tollerabilità della situazione. Ma quale tollerabilità, Ci dica quali sono i parametri di riferimento della tollerabilità. Forse pochi metri quadrati di una cella in cui sono stipati, in violazione dei più elementari diritti umani, i detenuti? Ci chiarisca perché, se le condizioni di tollerabilità delle strutture sono accettabili, un numero così elevato di ristretti si è suicidato o ha tentato il suicidio e perché direttori delle carceri, Polizia penitenziaria ed educatori hanno appoggiato le proteste perfino con scioperi della fame. Le condizioni delle carceri in Italia sono talmente inaccettabili che la Corte europea per i diritti dell'uomo, in occasione della sentenza 16 luglio 2009, in noto caso contro l'Italia, le ha espressamente dichiarate illegali. E tutto accade, come sottolinea l'appello dell'Associazione Antigone - Ristretti Orizzonti - Coordinamento nazionale dei Garanti dei detenuti, cui hanno aderito l'avvocatura, parte della magistratura e anche il Partito Democratico, nella pressoché totale disattenzione dei *media* e quindi dell'opinione pubblica, salvo ridestarsi nel periodo estivo, quando i palinsesti del circuito della comunicazione offrono un po' più di spazio e quando, con maggiore urgenza, si percepisce la drammaticità dei problemi. Ed è di questi giorni la notizia che il tribunale di sorveglianza di Lecce ha condannato l'amministrazione penitenziaria a risarcire il danno esistenziale provocato a un detenuto straniero, che sta scontando una condanna per furto, sottoposto ad una convivenza forzata con altri due detenuti in celle progettate per uno solo. Una situazione insostenibile, più volte denunciata e poi trasformata in numerosi ricorsi contro la condizione inumana e degradante della struttura. In effetti, i dati assoluti di sovraffollamento delle carceri, progressivamente crescenti, il numero dei suicidi e dei tentativi di suicidi dei detenuti, che denunziano una condizione di forte sofferenza umana, la percentuale dei detenuti in custodia cautelare, pari al 42 per cento, che esprime uno squilibrio in atto nel processo penale italiano, dimostrano la insostenibile drammaticità della situazione carceraria. E il Capo dello Stato ci ammonisce: «c'è un'emergenza assillante, dalle imprevedibili e al limite ingovernabili ricadute, che va affrontata senza trascurare i rimedi già prospettati e in parte già messi in atto, ma esaminando ancora con la massima attenzione ogni altro possibile intervento e non escludendo pregiudizialmente nessuna ipotesi. È evidente l'abisso che separa la realtà carceraria di oggi dal dettato costituzionale sulla funzione sulla funzione rieducatrice della pena e sui diritti e la dignità della persona; una realtà non giustificabile in nome della sicurezza, che ne viene più insidiata che garantita, e dalla quale non si può distogliere lo sguardo, arrendendosi all'obiettiva constatazione della complessità del problema e della lunghezza dei tempi necessari specie in carenza di risorse finanziarie adeguate - per l'apprestamento di soluzioni strutturali e gestionali idonee». Il Governo e il Parlamento, signor Ministro, non possono quindi sottrarsi al dovere di realizzare interventi strutturali che devono rispondere alla duplice esigenza di bloccare l'aumento del numero dei detenuti in ingresso e di avviare (appunto come ha auspicato il presidente della Cassazione, che anche lei ha richiamato nel suo intervento) un processo contrario teso ad una riduzione progressiva della popolazione carceraria. Noi, come Partito Democratico, non ci sottraiamo a un confronto. Siamo ben lieti di collaborare con lei. Siamo consapevoli che sia necessario approvare a breve, anzi a brevissimo, un progetto che punti alla riduzione della penalità e, in particolare della penalità carceraria, la cui espansione è frutto dell'aumento a dismisura della sfera del penale (altro che l'auspicato penale minimo!), espressione di un diritto securitario spesso irragionevole e teso verso una colpa d'autore (si pensi al reato di immigrazione clandestina su cui è intervenuta la Corte europea), dell'intensificazione della recidiva, dell'eliminazione e della restrizione di misure alternative. Lei ci dice, invece, che tra le cause del sovraffollamento vanno escluse, sia pure con molta prudenza, una particolare rilevanza delle norme introdotte nell'ultimo decennio a tutela della sicurezza. Delle due l'una: non si comprende l'utilità di tali interventi normativi in un'ottica di sicurezza; se poi non fosse giusta, come altri sostengono, occorre subito porvi rimedio. Se lei signor Ministro, intende veramente incidere sulla situazione delle carceri, occorre che faccia proprie (e oggi non l'ha fatto) proposte avanzate dal Partito Democratico in tale direzione: depenalizzazione dei reati minori; introduzione dell'istituto del non luogo a procedere per irrilevanza penale del fatto o la tenuità dell'offesa; sanzioni differenziate in ragione della gravità del reato, secondo i principi di sussidiarietà, offensività, colpevolezza; estensione agli adulti dell'istituto della messa alla prova. Sono tutti progetti, come dicevo, già presentati dall'opposizione, che possono essere rapidamente approvati in tempi brevi, ma ovviamente ben vengano anche disegni di legge del Governo, se questo può velocizzare l'*iter* di approvazione. Solo che lei oggi non ce li ha annunziati. Lei ci ha detto che meritano approfondimento l'attuale sistema della custodia cautelare e la disciplina dell' arresto facoltativo in flagranza. Ma noi pensiamo che ci voglia un cambio di passo, essendo convinti che occorre intervenire seriamente in materia di custodia cautelare

in custodia cautelare: ogni anno si registra il transito in carcere di 90.000 detenuti provenienti dalla libertà e di questi restano in carcere 21.093 fino a tre giorni, giorni, e 1.915 fino a sette giorni. Il carcere - sostiene il presidente degli avvocati delle camere penali - è una vasca che si riempie in continuazione a ogni emergenza sicurezza: occorre cancellare norme che impongono forme di custodia cautelare in carcere come quella della custodia obbligatoria ed evitare l'introduzione di norme nuove. Ed è questa, tra l'altro, la linea tracciata dalla Corte costituzionale, in particolare con una recentissima sentenza

chiarirci su alcuni interventi essenziali. Noi proponiamo, e lei non ce lo ha invece proposto oggi, un intervento sulla legge Fini-Giovanardi, che è causa di sovraffollamento. Inoltre, proponiamo un intervento sulla legge ex Cirielli, che ha contribuito in maniera esponenziale al sovraffollamento della carceri: come non porsi il problema dell'abrogazione delle norme che comportano aumento di pena in presenza della recidiva? Da ultimo, signor Ministro, lei oggi ci ha riferito sull'avanzamento del piano carceri. Noi riteniamo che siano informazioni importanti ma generiche, che non corrispondono ad una giusta esigenza dell'opposizione di conoscere con chiarezza, nel dettaglio, il programma di investimenti in edilizia carceraria. Non sappiamo nulla delle procedure di gara attivate e devo dire che più volte abbiamo rappresentato in questo ramo del Parlamento la nostra contrarietà a che al sistema carcerario si applicassero le norme della Protezione civile e che anche il direttore del DAP venisse a porsi, inutilmente, nella condizione in cui si è venuto a porre il Se quindi lei volesse apportare un cambiamento, noi saremmo ben felici di farlo. Sotto questo profilo, come già ha fatto il senatore Maritati, le confermo che siamo pronti a sederci a qualsiasi tavolo, purché si risolva questa situazione delle carceri e dei detenuti, che non è più accettabile in questo Paese.

che ci consentono di poter parlare - lo dico non per consolarmi, né per consolare il senatore Benedetti Valentini - a molte più persone di quelle che oggi possono apparire.

Ringrazio altresì, in modo particolare, il signor Ministro perché mi permette, per la terza volta, nel breve tempo dallo scorso novembre ad oggi, di intervenire su questo tema in quest'Aula con uno spirito di fiducia maggiore.

con grande attenzione. Abbiamo potuto rappresentare le scene drammatiche di una umanità ignorata e calpestata e abbiamo condiviso con tutta l'Assemblea la necessità che si intervenga, che questo sia un obbrobrio da superare.

Lo sa che non abbiamo saputo rispondere? Lo sa che ci siamo vergognati? Lo sa che non abbiamo avuto l'autorità sufficiente, quella che nasce dalla consapevolezza di un ruolo che si svolge appieno, per potergli rispondere? E io mi sono vergognato ancora di più perché sono anche medico.

di cui stiamo parlando in questo momento e a cui mi sto dedicando, hanno espresso parole di conforto e ravvisato una spinta significativa, per quello che oggi ci ha detto ed anche per il colloquio avuto precedentemente con il Presidente. È necessario riaprire questo discorso. Non possiamo continuare

mi vergognerei se ciò si dovesse dire di me e di noi. Signor Ministro, io ho fiducia che questo non lo si dica di nessuno di noi, proprio per gli impegni che ella oggi ha assunto, per quella sinergia che in qualche modo si sta strutturando tra le diverse parti dello Stato, perché è vero che sono solo 1.300 persone, ma lì c'è un disagio

più restare negli Opg! La riforma Basaglia, guardiamola come vogliamo, ma se inquadrata in quello spazio - lo dico agli uomini della destra che talvolta hanno potuto considerarla in modo diverso - è comunque estremamente positiva rispetto al degrado in cui queste persone sono state abbandonate.

per non poter presenziare ai loro interventi, che evidentemente leggerò domani sul Resoconto stenografico, ma purtroppo mi devo allontanare per un impegno di Governo correlato al Consiglio dei ministri di domani. Rivolgo a tutti loro le mie scuse.

Signora Presidente, non è sfuggita a nessuno la presenza costante, per tutta la giornata, del Ministro, per la quale lo ringraziamo. della prigione» è il titolo di un celebre libro di Michel Foucault, che introduce l'argomento del potere assoluto di fronte alla propria vittima giudiziaria. Damiens, imputato di aver tentato l'assassinio del re di Francia

Foucault parla dei corpi. Gli imputati sono corpi, non anime né intelletti. Il corpo è nella piena e totale disponibilità del potere assoluto. ci sentiamo lontanissimi da queste cose, però il discorso appassionato del senatore Saccomanno e la relazione

non ha quel totalitarismo intimo che era tipico del potere assoluto, però rappresenta un quadro di abiezione intima della società, incapace di porre un limite ad un diverso tipo

si compiace di restringere il condannato. O almeno così dovrebbe essere. Noi siamo tutti figli consapevoli e affratellati di una dimensione culturale che ci unifica tutti. Il condannato - l'imputato no, non dovrebbe nemmeno entrare in carcere, però ci entra ci entra - deve stare in carcere, quindi tutto quello che gli tocca è la restrizione. La Costituzione in materia è molto precisa: individua tutti gli gli atteggiamenti fondamentali con cui la giustizia deve prendersi cura dei suoi condannati. Stabilisce il principio della prassi rieducativa e del riavviamento alla società. alla società. Ma tutti noi sappiamo che i principi costituzionali sono spesso negati o opacizzati. Non c'è coerenza tra i principi severi e sobri, scritti con grande semplicità, della Costituzione e la prassi slabbrata, nascosta, omertosa e avvilita delle carceri italiane.

bisognerebbe arrivare all'improvviso e vedere cosa c'è. Il senatore Saccomanno l'ha fatto e ha raccontato in modo espressivo cosa può capitare di vedere in situazioni del genere. Non c'è solo la restrizione. Ci sono una quantità di violenze occulte e meno occulte; c'è la violenza della comunità incarcerata che si esercita all'interno di se stessa, di omicidi orribili (ricordo lo squartamento di Francis Turatello con un cucchiaio affilato, sventrato in un carcere sardo); c'è la violenza dovuta alla prassi di imposizione e soggezione sessuale nei confronti dei minori più indifesi; c'è la pura prevaricazione - ne ha parlato anche il Ministro in un passaggio - questa sorta di regime dove l'universo carcerato svolge una sorta di autosorveglianza e determina, dall'interno del carcere, all'interno delle leggi dello Stato, l'esercizio di sue proprie leggi, che hanno una cogenza forse maggiore (spazi che non si toccano, sguardi che non si alzano). Tutte cose che possono apparire soltanto psicologiche e che poi, invece, si traducono in morti volontari.

Chi avrà intascato i soldi per la costruzione di quel carcere inutile? Esattamente come chi sta intascando i soldi dell'inutile ponte di Messina, che non si farà mai e che però viene studiato e ristudiato.

non ci siamo. Voglio soltanto dire in questa sede che il quadro italiano è rigorosamente malato, perché la giustizia è stata inquinata all'origine

che insieme demoliscono in modo definitivo il processo penale, dovrebbe portare anche i colleghi pensosi della maggioranza a svolgere una riflessione autocritica. Potete davvero assistere, convinti di fare una cosa giusta, a questa sorta di sconcio di tutta la dimensione della giustizia italiana? In sostanza, la giustizia per l'uno - lo dico in modo ironico - e l'ingiustizia per tutti gli altri.

del Ministero della giustizia - ringrazio molto il garbo del Ministro e il Sottosegretario presente - si legge che il trasferimento delle funzioni sanitarie

quando attraverso un decreto legislativo fu deciso detto passaggio, ancorché ispirato a principi straordinariamente condivisibili, si pensò di aver fatto un grandissimo lavoro e che si trattasse di un passaggio di consegne. può invece scoprire che tutto ciò che serve per realizzare quel principio - tipo lo schema di convenzione per l'utilizzo dei locali tra le aziende sanitarie locali e le carceri, oppure i dati sanitari, i flussi informativi e le cartelle cliniche - è datato 29 aprile 2009. Questa è una piccola storia - a mio avviso - in cui ci si ritrova spesso, mi sembra riguardi il Parlamento: il fatto di enunciare spesso principi condivisibili e non riuscire poi ad arrivare ad enunciarli insieme con ciò che serve per farli vivere. Direi infatti che, per questa vicenda, è stato il cammino classico sul crinale, come quella squadra che, sapendo di dover cambiare allenatore e modulo, gioca

Sì, sono le carceri di quelle Regioni dove la sanità funziona bene. Ma noi sappiamo che 20 sistemi sanitari regionali stanno mettendo a dura prova quel diritto da esigere ugualmente per tutti ovunque. E mi pare che non vi sia dubbio che, là dove vi sono fragilità, questa esigenza diventa più complicata ancora. È evidente, che si riesce a dare con più difficoltà là dove le difficoltà aumentano, e mi sembra che le carceri rappresentino proprio quel luogo di fragilità. che questo ci debba servire in qualche modo anche da paradigma. Non si può certamente tornare indietro, e forse anche su questo una qualche accelerazione bisognerebbe darla. Ma sapere che,

Dopo l'intervento appassionato del collega Saccomanno e quello, più colto, del collega Pardi, mi avvio alla chiusura raccontando una piccola esperienza personale. Tra le finalità che hanno animato la necessità di passaggio della sanità carceraria dal Ministero della giustizia alle ASL c'era la promozione della salute Qualche anno fa (ne sono passati dieci)

nel mantenere la salute, rispetto alle difficoltà del quotidiano, fosse qualcosa che apparteneva più alla voglia del direttore di fare bella figura che non all'esigenza

Occuparmi della mia salute, cioè di non ammalarmi, mi ha dato un senso di libertà, come un anticipo di quando uscirò. Voglio una vita sana. Ho bisogno di stare bene e ho imparato da voi che si può fare e come si può fare. È una piccola contentezza di cui vi ringrazio. Qui dentro conta».

*(PD)*. Signora Presidente, ho chiesto la parola semplicemente perché mi ha molto allarmato l'intervento del collega, senatore Lauro, reso alla fine della seduta di ieri.

ci ha ricordato che, nel corso di questa legislatura, la Commissione antimafia ha approvato due relazioni sulle infiltrazioni mafiose nel gioco lecito e illecito: la prima nel 2009 e la seconda nel luglio del 2011. Ha dato anche una notizia veramente allarmante - ripeto - relativa all'uso del *web* per una serie di ammiccamenti alle fasce più deboli della popolazione, ai soggetti particolarmente a rischio, ai minori, in modo particolare, che sono letteralmente

A Lampedusa sono ormai mesi che si sta verificando una quotidiana e sistematica violazione dei diritti umani dei minori reclusi in una ex base militare

abbiamo cercato più volte, con un volo di linea, di recarci a Lampedusa, ma è tutto prenotato fino alla prima settimana di ottobre. Oggi la situazione si è aggravata ulteriormente, con gli scontri con la polizia che sono stati ricordati anche durante il nostro dibattito. Occorrerebbe capire dal ministro Maroni come intende affrontare la situazione. Abbiamo capito qual è la prima mossa, cioè quella dell'uso - abbastanza indiscriminato, mi viene da dire - della forza nei confronti di chi,

occorre capire se si tratta veramente di 7.000 nuovi posti o se è soltanto un gioco delle tre carte con cui si ripresenta alle Nazioni Unite il famoso piano di gestione dell'emergenza migrazioni dal Nord Africa. Occorre che il Ministro ce lo venga a dire, anche perché nelle prossime settimane ci saranno passaggi elettorali molto critici in quasi tutti i Paesi che hanno visto le cosiddette Primavere arabe. Non vorrei che, sulla scia di un aumento di questi arrivi, dovessimo ritrovarci qui, tra poche ore, ad adottare ulteriori nuove misure emergenziali che, come noi tutti sappiamo bene, non servono ad altro che a creare